Signor Presidente, onorevoli senatori, mi è stato chiesto di essere il più breve possibile, stante la dinamica dei lavori parlamentari di quest'oggi, e quindi di limitare al minimo le comunicazioni del Governo, allo scopo di ascoltare almeno parzialmente il dibattito parlamentare, in considerazione del fatto che l'appuntamento alla Camera è fissato tra meno di un'ora, in virtù dell'incontro di questo pomeriggio a Berlino con i *leader* di Germania e Francia. Dunque cercherò di essere il più breve possibile, contando sulla vostra comprensione rispetto alla sintesi della riflessione che sto per offrirvi. Molto chiaramente siamo di fronte ad una vicenda storica. Chi cercasse oggi di minimizzare o di strumentalizzare ciò che è avvenuto commetterebbe un errore politico di evidente rilievo. Il voto britannico sicuramente presenta caratteristiche anche di un qualche interesse per l'analisi sociologica e politologica britannica, ma è un voto che pesa come un macigno nella storia europea e come tale va considerato. Era già avvenuto quarantuno anni fa, nel 1975, ma il risultato era stato diverso.

Se passa il principio per cui il popolo vota e altrove si cerca di "mettere una pezza" su ciò che il popolo ha deciso, si mina alla base l'idea stessa del gioco democratico. Dunque, occorre questa consapevolezza, indipendentemente dalle opinioni da singolo. Questo mi sembra il primo punto. Non entro qui

Da parte nostra, credo che possiamo dire, come Italia, che tutto può fare l'Europa tranne che aprire adesso una discussione di un anno sulle procedure, dopo essere stati per un anno a discutere delle trattative. Se tutto è trattativa rispetto alle procedure, si perde di vista non soltanto il messaggio che arriva dal voto britannico, ma la stessa idea di Europa. Il primo tema quindi è che è accaduto qualcosa di enorme. *Ex malo bonum*, dicevano i latini. Credo che questo debba essere il nostro spirito. Le ragioni per le quali abbiamo criticato dall'interno le istituzioni europee, cercando di portare il nostro contributo perché le cose cambiassero, sono paradossalmente rese più forti che mai dall'espressione popolare britannica. E non soltanto per le dinamiche di quel voto, su cui non c'è tempo per insistere sebbene sarebbe molto interessante farlo. Mi riferisco in particolar modo al legame tra

per il *leave*. Come se l'Europa fosse divenuta, talvolta anche oltre le proprie responsabilità, il punto di riferimento di tutti gli scontenti. È un argomento sul quale dovremo ragionare e discutere nei prossimi mesi. Il punto centrale però è che se in questi mesi abbiamo chiesto un'Europa che fosse più sociale, che avesse a cuore l'immigrazione con uno sguardo onnicomprensivo, che si preoccupasse della generazione Erasmus, e fosse contemporaneamente capace di rassicurare chi appartiene ad un'altra generazione, se abbiamo fatto queste battaglie, le abbiamo fatte non perché volevamo affermare l'interesse dell'Italia - che pure ovviamente consideriamo un valore perché l'interesse nazionale è valore, non è disvalore nella discussione politica europea - ma perché ritenevamo che fosse l'interesse europeo, continentale e non soltanto l'interesse del nostro Paese. Dunque, a mio giudizio, quello che si apre domani è un vertice europeo, temo non sarà l'ultimo ad occuparsi di questi argomenti, ma che dovrà essere concentrato sul rilancio dell'Europa, non soltanto sulle procedure di uscita del Regno Unito. Dovrà essere concentrato su come reimpostare una strategia, sull'innovazione tecnologica, sull'artigianato e sui mondi vitali che possono essere nuovamente resi protagonisti da una strategia di innovazione tecnologica che non è contro la tradizione, ma è a sostegno della tradizione. Deve essere, a mio giudizio, questo il momento nel quale trarre insegnamento da ciò che è accaduto per riportare l'Europa alla sua forte identità. È l'Europa che combatte una battaglia di giustizia sociale e non soltanto una battaglia di procedure burocratiche. Da questo punto di vista, l'Italia è pronta a fare la sua parte. Noi abbiamo utilizzato l'espressione della «casa» perché essa non è soltanto un luogo fisico; per noi l'Europa è casa nostra. Io rispetto chi in quest'Assemblea, come alla Camera, ha da sempre espresso posizioni diverse. È un rispetto sincero che voglio rimanga agli atti. Nel senso che in quest'Assemblea ci sono famiglie politiche italiane ed europee che hanno opinioni diverse, non le hanno mai mandate a dire, hanno sempre avuto il coraggio della coerenza: c'è chi sta con la Le Pen, chi con Farage e chi con le famiglie tradizionali. Noi dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di prendere atto che questo può essere un momento di ripartenza se mettiamo al centro i valori che hanno fatto grande la nostra casa. La casa non è soltanto un luogo fisico, ma un luogo di sentimenti e di idee. Ecco perché abbiamo detto di ripartire da Ventotene e dalla formazione dei giovani ed ecco perché abbiamo chiesto di avere uno sguardo d'insieme globale che non fosse soltanto uno sguardo sull'orizzonte quotidiano, ma sul lungo periodo. Quello che però manca oggi è, a mio giudizio, la consapevolezza della gravità della situazione. Io non vorrei - e credo che questa sarà la linea con la quale noi ci avvieremo alla discussione - che si possa pensare di far finta di niente o che si possa semplicemente immaginare un percorso di riflessione molto, molto lungo, magari in attesa di un nuovo *referendum*. Tutto questo riguarda il Regno Unito; è una posizione che rispettiamo e ciò che decideranno i britannici sarà da noi rispettato fino in fondo. Ma quello che deve fare l'Europa oggi è smuoversi, perché se stiamo un altro anno ad aspettare che si ritorni sulle stesse regole su cui abbiamo discusso nell'ultimo anno, perdiamo l'appuntamento con le sfide e le priorità del nostro tempo. Guardate - e mio avvio rapidamente a concludere - cosa sta accadendo in queste ore in Europa e fuori: ci sono alcuni Paesi, penso alla Spagna, che tornano a votare e per la seconda volta nel giro di sei mesi non hanno un Paese governabile. Fa pensare il fatto che all'inizio di questa legislatura - l'abbiamo già detto anche in Senato - utilizzassimo tra di noi come un *benchmark* positivo il sistema spagnolo, perché fino ad oggi aveva dato Governi e governabilità chiara; non ce l'eravamo inventato quando ne discutevamo, era un dato di fatto. Oggi il sistema spagnolo, per la seconda volta nel giro di sei mesi, si trova al bivio: creare una coalizione di almeno tre dei quattro partiti, da quello che si vede, perché due potrebbero non bastare, oppure condannarsi alle terze elezioni nel giro di un anno. Quando si va a votare per due volte di fila nel giro di sei mesi cosa accade? I risultati non cambiano granché, ma la partecipazione sì, l'affluenza sì, perché viene meno il sentimento di fiducia nel gioco democratico. Pensate a quello che sta accadendo ‑ abbiamo discusso a lungo nel giudizio delle elezioni amministrative ‑ nelle periferie. Bene, parliamo delle periferie europee: lì sta il fronte più esposto della grande questione di sicurezza internazionale e nazionale. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire che non è respingendo l'idea di Europa che noi avremo più sicurezza, ma esattamente all'opposto: che settant'anni di pace stanno lì a dimostrare che l'Europa è forte se sta insieme, se è unita. Ma allora la cooperazione deve essere vera: sui temi della sicurezza, della difesa, sui fattori interni. Terzo e ultimo punto. Guardate che cosa accade fuori dall'Europa. Oggi - credo che sarà questione di ore - vi sarà l'annuncio ufficiale dell'accordo tra Israele e Turchia. Ciascuno di voi può avere le proprie opinioni; io ho appena discusso con il primo ministro Bibi Netanyahu a proposito di questo. È un segnale molto importante l'accordo tra Israele e Turchia, specie pensando a che cosa è accaduto negli ultimi dieci anni in quest'area geografica. Pensate a cosa sta accadendo al di fuori dei nostri confini. Abbiamo discusso più volte della Russia e dell'Africa. Il Consiglio europeo avrebbe dovuto avere al centro il grande tema del *migration compact*, portato dall'Italia per dare finalmente una strategia di lungo periodo sull'Africa e non soltanto un insieme di singole reazioni. Il mondo fuori di qui sta cambiando a una velocità impressionante. Permettetemi di dire che ciò che è avvenuto nel Regno Unito può essere la più grande occasione per l'Europa, se smettiamo di giocare sulla difensiva e se proviamo a dare al nostro Continente la possibilità di una nuova partenza. Perché questo accada, occorre buon senso ed equilibrio. L'Italia farà la sua parte, in tutti i i *format* che si renderanno necessari. Noi abbiamo sempre detto che il compito dell'Italia è quello di dare una mano, di costruire ponti e non muri. Per questo motivo abbiamo accolto l'invito a far parte oggi del tavolo a tre che discuterà a Berlino, con una novità. È un fatto inedito e al quale abbiamo dato l'adesione perché pensiamo che questo possa essere di aiuto, non perché cerchiamo chissà quale ruolo. Noi pensiamo che questo possa essere d'aiuto anche ai nostri amici francesi e tedeschi. Ma, accanto a questo, deve esserci chiara la direzione. La direzione non può essere quella di far finta di niente e di minimizzare. Il popolo britannico ha votato. Il voto vale, e questo voto ci impone di ripartire sull'Europa. L'Europa deve essere quella che si preoccupa un po' più di questioni sociali e un po' meno di questioni burocratiche. E accanto a questo deve esserci un'Europa dove le famiglie tradizionali, che hanno sempre detto di sì all'Europa, anche venendo da storie ed esperienze diverse, trovino in questo passaggio la grinta, la lucidità e l'intelligenza per capire che è il momento della responsabilità e non della improvvisazione; è il momento in cui tornare a credere in una Europa capace di suscitare speranze e non soltanto di generare paure.

Signor Presidente, la Brexit è stato un inutile esercizio di democrazia di un popolo che ha scambiato i suoi ricordi con il suo futuro? O, invece, come qualcuno ha osato dire, il popolo ignorante si è espresso e, siccome è ignorante, non può decidere su questioni complesse? In Italia lo dicevano già ai tempi del del popolo bue, definito da una cultura sessantottina che non accettava il volere della maggioranza. Quindi, i britannici ci rispondono ancora una volta con la celebre frase di Churchill, quella per cui la democrazia la democrazia è il peggior strumento di Governo, eccezion fatta per tutti gli altri che abbiamo verificato. O, invece, è piuttosto uno scacco alla regina Europa da parte di un popolo che di regine se ne intende e le ama. Un popolo che non perde una guerra da centinaia di anni. Lo schiaffo più umiliante, secondo noi, a un *establishment*, quello europeo, che ha divorato le democrazie europee. Lo ha potuto fare con la Grecia, ai tempi della Grexit; lo ha potuto fare con l'Italia, rovesciando un Governo eletto democraticamente con alchimie di Governi mai eletti dal popolo. Poteva farlo, secondo lei, con la democrazia più antica del mondo? No, soprattutto perché oggi siamo alle prese con il dramma della Brexit, esattamente come siamo stati prigionieri del dramma dello *spread* nel 2011 con la Grexit. I Paesi membri corrono a velocità divergenti, e questo vale non solo per l'eurozona, non soltanto per l'economia. Ma poteva dare lezione ai britannici un signore che, con la sua celebre frase «*out is out*» alla vigilia del voto, ci ha regalato questo bel risultato? Lui, il capo di un Granducato grande quanto una media Provincia italiana, che fa dell'evasione o, meglio, dell'elusione fiscale, che offre al mondo lo strumento del reddito suo e del suo Paese? È colpa di Cameron che, comunque, si è prontamente dimesso? O di Juncker, che ha dato il calcio finale a un'Europa messa in discussione per le tante ragioni che anche lei ha citato? Penso, ad esempio, alla questione dei migranti, con la gestione dei flussi e di quote di ripartizione dentro un *trend* demografico costantemente negativo, con una forbice preoccupante tra nuovi nati e nuovi sbarchi, che rischia di dare vita a una pericolosa equazione. Lo scollamento tra le istituzioni comunitarie e le istituzioni interne agli Stati è percezione comune, così come questa crisi economica mai davvero finita, le cui cause e meccanismi sono affari dei Governi centrali delle banche e del Governo comunitario, ma le cui ricadute

che oscilla tra la deregolamentazione e la sovraregolamentazione, creando cortocircuiti burocratici devastanti per l'economia. Ma è anche necessaria la riforma del regolamento di Dublino sull'immigrazione, tema discusso da molto tempo e da innumerevoli Consigli europei. Per non parlare poi della disoccupazione e di una comune lotta decisa contro il terrorismo, solo per citare alcuni dei grandi capitoli. Ecco che cosa c'è dietro Brexit: molto di più di una disputa sul modello economico e di una reazione arrabbiata, come taluni l'hanno definita. C'è il sintomo di un necessario e urgente cambio di passo che si impone. La ricetta c'è e passa anzitutto dalla rinegoziazione di tutti i trattati e di tutte le regole. Cambiare l'Europa, dall'interno, ma cambiarla davvero. Passare, per dirla con una formula breve e chiara, dalle costrizioni alla costruzione. Da tutte quelle imposizioni che ingabbiano gli Stati al rispetto di parametri e di *Diktat* che altro non fanno che che annichilire la vitalità economica e dei mercati interni ai confini nazionali, da un approccio punitivo fatto di sanzioni e di avvertimenti, a un'Europa che sappia invece agevolare autonomia e autodeterminazione, stimolare crescita e sviluppo, sostenere le imprese e muovere investimenti. Ecco da dove dobbiamo ripartire: da quel voto dei giovani contrapposti ai loro padri, che ci impone di riprendere la via che i fondatori dell'Europa definivano non facile, né sicura, ma che deve essere percorsa e che lo sarà: concludevano così gli autori del Manifesto di Ventotene che anche lei ha citato, signor Presidente. Forse più che rifarne un altro di manifesto basterebbe ripartire proprio da lì. Da quel «ce lo chiede l'Europa», a «ce lo impone l'Europa» a ricostruire l'Europa; ma lo potrà fare il suo Governo con pochi numeri, con poco consenso elettorale? Lo può fare lei, signor Presidente del Consiglio, che non ha saputo nemmeno utilizzare a favore dell'Italia l'azione forte e incisiva del governo britannico durante tutta la trattativa sulla Brexit? Era meglio fare squadra con chi metteva in discussione i meccanismi europei per un'Europa nuova, o fare l'anticamera per farsi accordare un po' di flessibilità sul *deficit* per mance elettorali e non per investimenti strutturali necessari al Paese? Lei l'ha avuta l'intuizione che per salvare l'Europa occorreva applicare a tutti gli Stati membri ciò che era stato riconosciuto al Regno Unito? E saprà opporsi alla prospettiva di un Ministro delle finanze unico europeo (ci manca solo questo!)? O invece, inseguendo il modello imposto della Germania, anche ai francesi, continueremo a scrivere direttive europee che i cittadini leggeranno come direttive tedesche? O farà fare all'intero Paese, signor Presidente del Consiglio, la fine che ha fatto fare alle banche italiane, ma soprattutto ai suoi risparmiatori, quei risparmiatori gabbati non tanto dalla crisi, ma da un Governo balbettante di fronte all'Unione Europea? Temo di no, signor Presidente, che lei noi ci riuscirà, e come me lo temono gli italiani, ai quali questo Governo prova a dire: «Dopo di me il diluvio. State attenti», perché gli italiani stanno già rispondendo che probabilmente il diluvio è proprio questo Governo.

Quindi ben venga il voto degli altri ma il nostro voto, il voto dei nostri concittadini non viene neanche preso in considerazione, come se fossimo in una monarchia. la società che fa da euro-barometro, che analizza il polso dei cittadini europei, ci dice molto chiaramente, nell'ultimo sondaggio, che solamente il 49 per cento degli italiani è a favore dell'euro e di conseguenza siamo la Nazione europea con l'indice più basso. Ci sarebbe piaciuto capire, e capire insieme, che cosa ne pensano i nostri concittadini.

Europa le servisse per risolvere i problemi sul fronte interno. Quindi i suoi interlocutori (non noi, non Farage e non la signora Le Pen, i suoi interlocutori - ripeto - già mettono in dubbio l'autorevolezza della sua presenza in Europa.

che il fronte del *leave* fosse forte in Europa perché l'Europa non è considerata dai cittadini britannici un interlocutore in materia di lotta all'immigrazione. Ricordiamo, Presidente, Frontex, Mare sicuro, Euformed, tutte iniziative della sua Europa, della vostra Europa che hanno solamente lo scopo di fare da raccoglitore e traghetto di migranti. A cosa sono servite, Presidente, queste missioni? A nulla. Queste missioni non sono servite a nulla. Sono servite solo ai cittadini europei per essere sempre più consapevoli come anche sul tema dell'immigrazione l'Europa non stia facendo nulla perché l'Europol dichiara che nel 2015 i trafficanti di esseri umani hanno guadagnato, grazie a questo traffico, tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Di conseguenza che cosa sta facendo l'Europa e cosa sta facendo l'Italia? Non stanno facendo nulla. E l'Italia prima su tutti. Quindi, le chiedo di partecipare al Non sta facendo deterrenza perché nei Paesi africani la nostra Marina militare viene vista un po' come un traghetto: miliardi e miliardi di euro di navi della Marina militare, ministro Pinotti, vengono utilizzati come la MSC o come la Costa Crociere. Utilizziamole per fare Non abbiamo credibilità militare, anche in questo caso a livello mondiale: spendiamo 1,27 miliardi di euro in missioni all'estero, mandiamo i nostri bersaglieri in Iraq e in Afghanistan ma non si sa a fare cosa.

Le chiediamo, signor Presidente del Consiglio, di parlare di lavoro e di tutte le problematiche che affliggono i cittadini europei, ma soprattutto i cittadini italiani. Le chiediamo anche, visto che qualche giorno fa lei è stato a San Pietroburgo e ha parlato con il presidente Putin, di andare in Europa e di far sì che la Russia non sia l'unico problema della sicurezza a livello internazionale, perché è quello che sta dicendo in questo momento la NATO. Noi chiediamo che le sanzioni alla Russia vengano tolte; chiediamo

è casa sua e di quella parte degli italiani che la reputano Europa; ma questa Europa non è casa mia. Io non sono uno dei giovani che ha fatto l'Erasmus, ma sono uno di quei giovani che negli anni Novanta faceva l'Interrail, quindi l'Europa la conosce bene. Dopo dieci Interrail posso dirle che questa Europa non mi piace: preferivo l'Europa delle Nazioni e dei popoli, anziché quest'Europa delle sue amiche banche e dei suoi amici poteri forti*. Signor Presidente, signori senatori, i fatti di questi giorni ci dimostrano, in modo drammatico, la centralità della questione europea. Certo, l'Europa è già entrata - e in vasta misura - nella nostra vita. L'80 per cento della legislazione interna italiana, ad esempio, è già di matrice europea. Si va dalle materie più importanti (si pensi, ad esempio, alla materia del risparmio) per arrivare a quelle più stravaganti. A titolo indicativo, ancora due mesi fa in questa sede si votava una legge comunitaria che si occupava imperterrita di basilico, di rosmarino, di salvia e di tartufi. Ma, certo, la centralità della questione europea emerge oggi, in forma assoluta e drammatica con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. A fronte della crisi, lei, signor Presidente del Consiglio, ha detto che la sua visione, la sua azione e, soprattutto, la sua nuova Costituzione sono fatte per difenderci. Ci si permetta di dubitarne, soprattutto di quest'ultima. Sul quadrante europeo la nuova Costituzione non è, infatti, e non sarà affatto, uno scudo protettivo, ma piuttosto un pericolo aggiuntivo. Nella storia, nel mondo, non c'è il caso di una Camera, quale sarebbe il nuovo Senato, con origine locale ma con competenza internazionale e, in specie, con competenza proiettata su una materia strategica e decisiva come soprattutto oggi è quella europea. Materia su cui, tanto per restare nell'Unione, quanto per uscirne, comunque ruota e ruoterà di qui in avanti l'asse della politica di tutti gli Stati europei. La nuova Costituzione italiana sarebbe un male in tempi normali, ma sarà un tragico errore nel tempo di ferro che sta arrivando. Negli articoli 55 e 70 si parla quattro volte di Unione europea, per dare al nuovo Senato competenza legislativa concorrente e paritetica, in un caso esclusiva, in materia di rapporti dell'Italia con l'Unione europea. A chiusura, nell'articolo 87, si dispone che il Presidente della Repubblica: ratifica i Trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione previa autorizzazione delle Camere, cioè di entrambe le Camere.

addendi eterogenei che avranno competenza sul rapporto dell'Italia con l'Europa e perciò competenza sul nostro destino. Saranno forse politici meno numerosi, ma molto più potenti di prima in una compagine che, via, via, fatalmente sarà diversa da quella che forma la maggioranza politica della Camera, sempre più eterogenea, casuale, erratica, dotata di un crescente potere di voto, di veto e di ricatto. Più di due anni fa, signor Presidente, lei è venuto per la prima volta in quest'Aula annunziandosi come l'ultimo Presidente a chiedere la fiducia al Senato. Da ottobre potrebbe avere ragione per pentirsene dovendo recarsi nel suo nuovo Senato, un Senato vischioso e paludoso, per chiedere voti sempre più decisivi per le sorti del Paese, ma senza poter imporre la fiducia.

è stato concentrato, distorto: un bicameralismo suicida. Una Costituzione, la sua, che non porterà la fine della confusione, ma piuttosto una confusione senza fine. Si noti per inciso che chi semina *referendum*, non necessariamente raccoglie plebisciti. Quello del Regno Unito è l'incidente del futuro: per fortuna, si è verificato ancora prima che la Costituzione entrasse in funzione. Potremmo dire che non è stata colpa di nessuno ma su questo, almeno per una volta, nell'interesse del Paese, ascoltateci! Ciò premesso, e se ci è permesso, ancora da questo vecchio Senato guardiamo all'Europa e allo «Stato dell'Unione». Altre volte, anche in questa Aula, abbiamo avvertito sull'arrivo di una crisi generale dell'Europa. Lo abbiamo fatto notando come negli ultimi vent'anni in Europa e sull'Europa si siano via via addensati ma siano stati festeggiati, del tutto ignorandone il lato oscuro - in sequenza quattro principali fattori di crisi: l'allargamento; la globalizzazione; l'euro; l'assenza nei Trattati dell'ipotesi che una crisi potesse arrivare. Come se il bene fosse la regola ed il male invece l'impossibile. E poi ancora le migrazioni e la distruzione del lavoro causate dalla rivoluzione digitale. molti sonnambuli continuano a credere che, tutto sommato, si sia ancora nel «migliore dei mondi possibili»; che non ci siano stati da parte loro errori o colpe, semmai solo errori o colpe da parte dei popoli; dominante ancora l'idea che siano i governanti a poter scegliere i popoli e non i popoli a scegliere i governanti. Tutto in realtà è cambiato e non si può continuare a credere che sia sufficiente fare quanto si sta facendo: il lancio di interdetti e di esorcismi, la demonizzazione dei popoli, condannati come autori di inammissibili secessioni della plebe; l'aggiornamento delle *family photo*, semmai solo con qualche sbianchettamento; la stesura di dichiarazioni e comunicati congiunti di impegno, che in realtà dimostrano più debolezza che forza; l'invenzione di nuovi tipi di direttorio, per esempio, l'ultimo sarebbe fatto a *troika*. A chi considera un successo l'entrarci, va ricordato che il lato giusto della storia non è più al vertice, ma alla base. È sempre più chiaro che non si possono gestire fenomeni così forti e così nuovi con formule che sono tanto vecchie quanto sbagliate. Dunque, abbiamo davanti tre ipotesi principali: la prima, continuare a credere che possa ancora reggere una Unione sopra gli Stati; una Unione che pretende di avere e ancora di conservare - potere senza responsabilità sopra, e senza democrazia sotto: liberi tutti di parlare e di votare su tutto, su tutto, tranne che sull'Europa! Secondo scenario: ritornare a Stati tra loro isolati, padroni del loro passato, ma fatalmente destinati ad essere dominati da forze globali che si sono già viste essere ancora peggiori di questa Europa. Non si può certo escludere che si arrivi a questo passaggio, ma, prima che sia così, abbiamo un dovere politico e storico, il dovere di provare a tornare allo spirito creatore dell'Europa, come era negli ideali originari e come poi è stato invece tradito, sovvertendo la regola costituzionale fondamentale della sussidiarietà nel rapporto tra gli Stati e l'Unione europea. Noto che su questo punto essenziale molto saggiamente si è pronunciato, nei giorni scorsi, il presidente Berlusconi. Terzo scenario: non una Unione senza gli Stati, non Stati senza Unione, ma sostituire i vecchi Trattati con nuovi «articoli di confederazione». Farlo a partire dagli Stati nazionali, che non sono più, come mezzo secolo fa, pericolosi incubatori di guerre, ma provvidenziali contenitori di quel che resta della democrazia. Su queste basi, riscrivere i Trattati *ex novo*, definendo cosa può essere fatto meglio sopra, a partire, per esempio, dalla difesa, ma lasciare sotto tutto il resto, come è appunto nella logica e nel principio della sussidiarietà. I popoli sono più saggi di Bruxelles nello scrivere le leggi destinate a governare la loro vita nella libertà e per la prosperità, senza alcun bisogno del dominante integralismo giuridico europeo. In conclusione, tra insistere su di una utopia fallita e perciò senza futuro o tornare ad un passato forse pure questo senza futuro, occorre invece cercare, almeno per un'ultima volta, di far prevalere l'ordine sul disordine e la ragione sulla follia. Sono infatti gli Stati nazionali e sono i loro popoli che, confederati nella libertà e nella democrazia, oggi hanno ancora l'onore e l'onere di alzare in Europa la bandiera della civiltà occidentale. È solo così che si può aprire la strada verso un futuro che sia migliore del presente: un futuro che abbia ad essere migliore per noi e per i nostri figli. Signor Presidente, il *referendum* in Gran Bretagna è stato uno *choc* per l'Europa, ma gli squilibri dell'Unione sarebbero rimasti intatti anche se i britannici avessero bocciato le spinte euroscettiche. Ora bisogna andare avanti e io credo, Presidente, che non sia un'eresia definire il nostro *referendum* d'autunno sulla riforma costituzionale come un passaggio altrettanto cruciale di quello britannico, non solo in chiave italiana, con la da lei preannunciata "Renzit" in caso di vittoria del no, ma anche e soprattutto perché una sconfitta delle riforme ci farebbe compiere un gigantesco salto all'indietro sul fronte della credibilità nell'Unione Sarà quindi un *referendum* sulla stabilità dell'Italia, nel bel mezzo della tempesta perfetta in cui si trova l'Europa, tra flussi migratori in aumento, crisi demografica, rischio terrorismo, instabilità dei mercati, fragilità delle banche, incertezza sul debito ed economia in stallo, con le conseguenti pulsioni antisistema. Dunque, la bocciatura di una riforma attesa ormai da decenni aprirebbe una crisi politica gravissima, un Parlamento delegittimato dai cittadini dovrebbe esprimere non si sa quale Governo e sarebbe arduo perfino tornare alle urne senza una legge elettorale coerente. L'Italia ha riacquistato credito in Europa e sui mercati promettendo e attuando riforme strutturali. Se non passasse la madre di tutte le riforme, quasi certamente alla crisi politica si aggiungerebbe una crisi finanziaria anch'essa gravissima.

ma attualmente è una casa in fiamme, e in questa situazione l'Italia non può permettersi di lasciare campo libero agli avventurismi, al tanto peggio tanto meglio, È una consapevolezza che dovrebbe accomunare tutte le forze che si riconoscono nei grandi partiti che hanno fondato l'Unione europea. La domanda ineludibile da porsi, però, è se prima che la Gran Bretagna uscisse dall'Europa non sia stata l'Europa ad uscire da se stessa, tradendo con la deriva finanziaria e burocratica quella che per mezzo secolo aveva garantito pace e prosperità. Ora siamo ad un bivio cruciale e le opzioni possibili sono essenzialmente due: più integrazione alla Schäuble, e dunque una maggiore disciplina finanziaria, oppure più concessioni in materia di bilanci, fisco e banche. Su questo fronte è giusto riconoscere che l'Italia è in parte riuscita a cambiare verso all'Unione, spingendola dal rigore a senso unico della Germania all'opzione prevalente della crescita. Ma dal *fiscal compact* al *bail in*, i danni sono già stati ampiamente fatti. Ci vuole un compromesso fra le due opzioni, partendo però dal dato reale che in questa lunga crisi la Germania si è presa troppi privilegi a scapito di tutti gli altri, ben oltre il dettato del primo Trattato di Maastricht, che non prevedeva piani di rientro a tappe forzate. La storia di questi anni ha già dimostrato che in un'unione monetaria, il *surplus* di un Paese produce più danni dell'eccesso di *deficit* di altre economie e che abdicare al controllo dei confini esterni non può non creare sconcerto, insicurezza e rigetto in ampie fasce della popolazione. Su quest'ultimo punto, va detto che il *dossier* sull'immigrazione è stato ed è un fallimento totale ed è inutile sostenere che l'immigrazione da problema italiano è diventato un problema europeo, perché non è vero. La Commissione europea non è infatti riuscita a indirizzare gli Stati membri verso una politica migratoria comune, mettendo così potenzialmente in discussione sia la validità di Schengen, sia la realizzazione del sistema comune di asilo europeo che superi una volta per tutte il Regolamento di Dublino. L'Italia ha fatto il suo dovere salvando migliaia di vite nel Mediterraneo, ma l'Europa ci ha lasciati soli: abbiamo almeno il coraggio di dirlo senza rivendicare successi che l'opinione pubblica non vede e non sente. Anche da questo, dalla capacità del Governo di farsi sentire autorevolmente in Europa, dipenderà l'esito del *referendum* cruciale di ottobre.

più chiare rispetto alla posizione che il nostro Paese assumerà domani, durante il vertice europeo e anche nel ristretto vertice di oggi pomeriggio a Berlino, perché intanto dobbiamo avere la consapevolezza di un'analisi seria del voto in Gran Bretagna. Lo dico qui in modo molto chiaro: noi non riteniamo assolutamente convincenti alcune letture che sono state date, tipo quella del conflitto generazionale, e i dati ci confortano in questo senso.

Questo voto ribadisce con chiarezza la sfiducia ormai di milioni di cittadini europei nei confronti delle politiche europee, del rigore e dell'*austerity*, sfiducia che diventa una vera e propria rabbia popolare

in una situazione in cui alla crisi economica non sono state date risposte adeguate, che pure erano necessarie;

quindi di uno dei fattori che storicamente ha rappresentato un elemento di stabilità in tutti i nostri Paesi. Non c'è sfiducia solo nei confronti delle politiche europee, ma anche, in generale, nei confronti della politica come strumento per poter cambiare la propria vita, perché si ritiene che, di fronte ai problemi dei cittadini colpiti dalla crisi,

Tutti noi siamo legati al Manifesto di Ventotene e ai valori dell'Europa, ma oggi non basta più, non è sufficiente fare solo e unicamente questo richiamo.

Non ci si può accontentare di essere stati invitati nel salotto buono, perché la foto che ritrae insieme Renzi, Merkel e Hollande rischia di essere una cartolina sbiadita che non avrà

affrontare con forza e in modo definitivo la revisione del *fiscal compact.* Tutte le nostre politiche in quello spazio di sovranità nazionale che era rimasto, alla fine sono andate sempre in quel senso.

per dire questo, vi state incamminando su una strada sbagliata. E ve ne accorgerete, perché i cittadini quando votano, come vedete, danno segnali chiari e precisi.

Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, in questo tornante della storia si concentrano eventi che concorrono tutti ad alimentare processi di disgregazione nelle comunità tra nazioni e nelle nazioni stesse. Coloro che si percepiscono come perdenti nella nuova dimensione globalizzata pensano di essere in balia di un mondo senza guida, sperano nella rottura dei vecchi assetti, perché credono di non avere null'altro da perdere che le proprie catene, cercano rifugio nella ricostruzione di un'autosufficiente (o quasi tale) sovranità nazionale. Il Presidente del Consiglio ha opposto a questi processi una fase di responsabilità e di riforme in Europa, cui dovrebbero concorrere in primo luogo le due tradizionali famiglie politiche, ripartendo dai valori depositati dalla storia comune; valori che nei Trattati furono invero negati, nel nome di quel relativismo culturale che ci ha reso tutti più fragili. Ma la costruzione responsabile di un migliore futuro europeo non può prescindere dalla dimensione nazionale e dalla ricomposizione in essa di una parte almeno dei molti processi di disgregazione. Tanto più che la nuova Europa si potrà ragionevolmente definire sulla sola base che allo stato appare sostenibile, quella confederale. È l'ora insomma, anche in Italia, di una fase di responsabilità repubblicana, che impegni in primo luogo il Governo ad iniziative di apertura nei confronti di tutte le opposizioni, affinché si possano condividere almeno i profili fondamentali dei nuovi assetti istituzionali interni ed europei, perché tutti possano sentirsi a loro agio e più sicuri Signor Presidente del Consiglio, lei disponeva di una maggioranza parlamentare a sostegno del suo Governo e di una più larga maggioranza a sostegno della riforma costituzionale. La seconda avrebbe dovuto naturalmente condividere la scelta della prima carica dello Stato e la legge elettorale. Il gioco delle maggioranze variabili, che lei ha preferito, si è risolto in una profonda divisione rispetto non solo alle politiche pubbliche, ma alle stesse regole del gioco democratico. Vi è stata poi recentemente l'opportunità di dare una risposta pragmatica e condivisa alla domanda di diritti certi da parte delle stabili convivenze omo ed eterosessuali, ma, com'è noto, si è preferita una soluzione ideologica in favore della famiglia artificiale, lacerando la nazione su ciò che in termini di principio e di concreta esperienza più l'ha formata. Non insista lungo questa via e si apra alla paziente ricerca di una base condivisa sui grandi capitoli della nuova Europa, così da ottenere ai tavoli della negoziazione quell'ascolto che meritano gli autentici *leader*, quelli che sanno essere inclusivi. Penso in particolare al rapporto tra la sovranità nazionale e i poteri europei, ai termini dell'unione fiscale e bancaria, alle politiche di sicurezza per la gestione della pressione migratoria e delle instabilità che la generano. Ma come proseguire nel frattempo lungo la via che conduce ad una scadenza referendaria lacerante? Non sarebbe impossibile avvicinare le posizioni sulla stessa legge costituzionale, se si aprisse un confronto sincero sulla riforma elettorale, che ne costituisce complemento dirimente, e sulle leggi di attuazione che dovranno regolare i nuovi contrappesi alla semplificazione e concentrazione del potere democratico. L'esperienza di questi mesi ha insegnato che la stessa crescita interna, condizionata oltretutto dalla depressione del commercio globale, non si genera soltanto attraverso politiche di incoraggiamento, pur necessarie, degli investimenti esteri o una migliore regolazione tarata sulle imprese più strutturate. Una nuova stagione di sviluppo italiano si può produrre solo da una mobilitazione diffusa della nostra comunità, da quel capitalismo popolare e familiare che nei servizi o nelle manifatture trasformate dalle tecnologie digitali può ancora generare lavoro e ricchezza. nulla più della coesione nazionale, del sentirci parte di un comune destino, può dare luogo a questa mobilitazione. Sia lei per primo inclusivo e aperto all'ascolto e forse, in luogo del circolo vizioso che sta esaltando tutto ciò che ci divide, si aprirà il circolo virtuoso che fa riconoscere ciò che ci unisce. Per il bene di tutti, soprattutto dei più deboli. Governo, innanzitutto vorrei che rimanesse a verbale il fatto che questa giornata è stata abbastanza complicata sotto il punto di vista organizzativo e, al momento, neanche sappiamo chi ci risponderà in Assemblea. Probabilmente il Il presidente Renzi ha iniziato il suo discorso dicendo che un macigno si è abbattuto sull'Europa.

più volte dicendo, ad esempio, che le scorse elezioni amministrative erano un fatto locale e non potevano avere riflessi sul Governo centrale. centrale. Allo stesso modo, questa mattina ci ha detto che l'esito del *referendum* nel Regno Unito è un fenomeno globale che probabilmente non avrà effetti, neanche questo, sul Governo italiano.

In effetti, quello che è successo in passato non ha mai avuto effetti sul Governo Renzi e faccio qualche esempio: Mafia Capitale non ha determinato neanche uno scossone sul governo Renzi. Piazzare degli emendamenti ad uso e consumo delle *lobby* del petrolio non ha avuto ripercussioni sul Governo; avere due morti italiani in Libia non ha avuto ripercussioni sul Governo; un giovane italiano massacrato in Egitto non ha ripercussioni sul Governo; favorire le banche e mandare sul lastrico i risparmiatori italiani non ha un effetto su questo Governo. Mi chiedo allora: secondo voi, cosa ha un effetto diretto su questo Governo? O siete in un delirio di onnipotenza? In realtà,

parlano di popoli differenti, ma il risultato è semplicemente lo stesso, perché parla degli effetti delle vostre politiche. Ci state mettendo l'uno contro l'altro; uomini contro donne, periferie contro centro, privilegio contro sacrificio. È questa la politica che state mettendo in atto ed è quella che vi ha portato I punti in comune, invece, tra Renzi e Cameron sono molti. Uno tra tutti: Cameron è stato travolto da un *referendum* che egli stesso ha voluto e, probabilmente, sarà anche l'esito del *referendum* che voi stessi state chiamando Il fallimento sta anche nel fatto che quello che proponete voi, tiranni europei, è un'Unione europea a trazione sostanzialmente finanziaria: tagli ai servizi pubblici, tagli agli enti locali e alla sicurezza lavorativa, ma soprattutto ripianamento dei bilanci sofferenti delle banche, soffocando il tessuto industriale delle piccole e medie imprese italiane. Tutto questo senza mettere in discussione, neanche una volta, i Trattati, che non sono mai stati discussi e ratificati dai cittadini italiani. Come farà questo Governo, con un PIL meno forte del previsto, a rispettare le sue promesse nel 2017 e ad evitare che scattino le clausole di salvaguardia, con l'ulteriore aumento dell'IVA? Sarà impossibile, se non approvando altri tagli, che andranno ad incidere sulla carne viva degli italiani. È questo il vostro piano, a questo servono le riforme costituzionali: a trasformarvi nei procuratori fallimentari dell'Italia. Austerità, trattati insostenibili, disoccupazione e stagnazione. Questa è l'Unione europea che lei accetta da quando è al Governo, nonostante faccia finta di combattere con il coltello tra i denti. Lei, presidente Renzi, non ha ottenuto un centesimo di quello che il Regno Unito otterrà grazie al *referendum* richiesto dal Primo ministro, e che in parte aveva già ottenuto prima del *referendum* perché stiamo parlando di un Paese, il Regno Unito, che già non aveva l'euro e non rispettava trattati quali il *fiscal compact*. Concludo questo intervento suggerendo due mandati principali per questo pomeriggio. Il primo: i cittadini britannici si sono già espressi ed hanno scelto, quindi l'Italia dovrebbe sostenere questa decisione democratica e assecondare le decisioni prese dal popolo Purtroppo, lei e questo Governo non credete nella democrazia e nelle decisioni del popolo, ma credete soltanto in voi stessi. E poi un secondo mandato: che dobbiamo fare in modo che l'Europa sia la nostra casa. Questo pomeriggio, mentre sarà in Europa a fare merenda con gli altri tiranni europei, dovrebbe dire agli altri tiranni europei che se casa deve essere, gli italiani vogliono le chiavi di quella casa. Perché ci sono soltanto due possibilità in cui una persona sta in una casa e non ha le chiavi: o è un adolescente o lo hanno rapito. Siccome il presidente Renzi mi sembra che entri ed esca con molta disinvoltura da tutte le porte, probabilmente è vero il primo caso. dico, allora: smetta di essere adolescente, vada in Europa e tuteli gli interessi dei cittadini italiani, di tutti i cittadini italiani, non soltanto di quelli che pagano le campagne elettorali.

del Governo, non vi è dubbio che il 23 giugno segni una data simbolica per la storia d'Europa; è un atto politico, così va letto, e come tale chiede una risposta politica. Tra le molte difficoltà che provoca, vanno cercate anche, come ha sostenuto il Presidente del Consiglio, le occasioni e le opportunità che presenta. Intanto, per l'immediato, ciò che è accaduto riequilibra la gerarchia dei problemi che è urgente affrontare. Ci consente, ad esempio, qui oggi, di allontanarci per un momento dal finto dramma del cambio di domicilio di qualche Sindaco, per metterci davanti alle vere grandi sfide che cittadini e popoli sono chiamati ad affrontare. Un breve cenno a un problema enorme, che non possiamo qui approfondire, ma cui andrebbe dedicato molto e intenso pensiero politico. Appunto, cittadini e popoli. Si è creata una sorta di discrasia, una contraddizione tra queste due dimensioni del vivere pubblico, insopportabile per un sistema democratico. La cittadinanza non si riconosce nella nazionalità, tende ad arretrare in soluzioni localistiche, particolaristiche, diciamo pure privatistiche. Il rischio dell'effetto domino non riguarda tanto la possibile uscita di altri Paesi, pur presente, quanto all'interno di alcuni Paesi la ripresa di rivendicazioni autonomistiche. Il voto vede divisi inglesi, irlandesi, scozzesi, gallesi e, magari, londinesi. Ci sono delle condizioni oggettive per questo: c'è il fenomeno dell'immigrazione di massa che impatta con il disagio sociale crescente provocato dalla crisi economica e crea differenti approdi, approdi, che fanno emergere uno stato di malessere, anch'esso di natura e di sostanza politica. il problema dell'Europa. Come si fa a predicare sovranazionalità in un momento che vede un arretramento di opinione al di qua della stessa nazione? Per l'idea che mi sono fatto della politica, in questi casi non bisogna inseguire i processi, non semplicemente rappresentarli, ma contrastarli, fino a rovesciarli. Questo è ciò che distingue una grande forza politica, armata soggettivamente di un progetto, con vera responsabilità di Governo che guarda, come è stato detto, non alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni, e la distingue da piccole formazioni minoritarie, il cui unico programma è quello di lucrare su una contingenza magari, favorevole. Penso anch'io che esistano i bisogni vitali ed essenziali delle persone (lavoro, immigrazione, sicurezza), che vanno posti avanti a tutto, ma che vanno essi stessi già inquadrati in un progetto di rilancio dell'unità politica. Mostrare, e dimostrare, che una crescita economica comune viene facilitata dal farsi, da parte dei cittadini delle nazioni, un popolo europeo. Più ancora che cittadini europei, quindi, popolo d'Europa. Questa economia di crescita comune, sul modello di un'economia sociale di mercato, da molto da molto tempo dimenticata, è il punto dove il sociale cerca di mediare ed arriva a mediare, tra economia reale da una parte e mercati finanziari dall'altra. La sentenza emessa il 23 giugno recita: non colpa delle masse, ma fallimento delle *élite*. Si è lasciato consumare, fino a spegnersi, quell'ideale che l'età dei fondatori europeisti aveva messo all'ordine del giorno dopo le tragedie del Novecento. Le ha richiamate, queste personalità, il nostro presidente Napolitano nell'introdurre alcuni suoi interventi sul tema. Non a caso, intitolava il libro: «Europa, politica e passione». Passione, appunto. Il compito della politica è oggi quello di risvegliare questa passione per l'Europa: sapendo realisticamente che viviamo nel tempo di tutte le passioni spente. Ma appunto per questo, bisognerebbe mirare alla formazione di una classe politica di stampo neoeuropeo, con il compito di sollevare questo tempo incerto ad una dignità d'epoca. Se esistesse un partito del socialismo europeo farebbe di questo la sua missione storica. Ci vorrebbero nuovi Ci vorrebbero nuovi profeti ad infiammare i popoli: unico antidoto, questo, a che i cittadini, appunto, vengano infiammati, al contrario, da improbabili, improvvisati, irresponsabili demagoghi, che rischiano ora di avere libero campo. Problema: come fare in modo che questo che attualmente appare, ed è, realmente, un sogno, cominci a realizzarsi praticamente? Di questo si deve parlare. È necessario, certo, che vengano fatti piccoli passi, ma tra i piccoli passi inserire momenti e scatti di accelerazione e di anticipazione. Un primo passaggio potrebbe essere questo. Affinché nei singoli Stati ritorni il primato, perduto, della politica, occorre che i singoli Stati tornino a praticare il primato della politica estera. Ecco uno dei punti su cui centrare il discorso. Nell'età della globalizzazione economica, globalizzazione economica senza politica, fare sì che la politica estera diventi una obbligazione statuale. ci ha spiegato che le democrazie non sono in grado di mantenere una politica estera di lungo respiro. È ovvio perché: perché di breve durata sono i Governi e di facile mutazione l'opinione da cui elettoralmente dipendono. Pensate, per fare un esempio decisivo, alla differenza di gestione delle questioni internazionali tra un George Bush e un Barack Obama, pensate all'abisso che si potrebbe creare tra un Obama e, Dio ce me scampi, un Trump. Ma non è questo il punto. Il punto è come impiantare una politica estera di rango europeo, almeno sul medio periodo. Il compito immediato è uscire al più presto, con tutti i mezzi, dall'emergenza terrorismo, con tutte le conseguenze che sappiamo provoca, per riacquistare lungimiranza di movimento, che ci viene impedita da questa emergenza. Non riusciamo a pensare all'Europa di domani, circondati come siamo da quello che ribolle ai nostri confini e di riflesso anche dentro i nostri confini. Dopo, e nel frattempo, che fare? Esprimo un'idea che so molto controversa attira molte controrepliche nella condizione storica attuale. Ma cerco - e credo dobbiamo cercare insieme - una via di uscita dallo stallo in cui si trova l'idea politica di Europa. Insomma, questa Europa è oggi un treno con tanti vagoni. Forse, troppi. L'allargamento - si sta riconoscendo da varie parti - non è stato ben ponderato. Risulta assai squilibrato:

Siamo di fronte qui a una sorta di *handicap*, non immediatamente rimediabile, ma che resta lì come grande problema irrisolto. La realtà è che i vagoni da soli non camminano. I mercati li fanno girare intorno a se stessi, ognuno per suo conto. Ci vuole una locomotiva politica che li traini verso una direzione precisa. Una Unione a due velocità economiche, si dice; sì, ma anche a due velocità, una economica, una politica. Un'Unione economica larga e un'Unione politica stretta. Questo nuovo e antico Centro-Europa - mi lascio guidare da tutte le mie nostalgie culturali mitteleuropee - ha già un centro, storico-naturale, ed è la Germania. Questa immagine della Germania ridotta allo spauracchio dell'*austerity* è di corto respiro. Francamente, a questo punto, preferisco un asse tedesco a un asse francotedesco. Intorno a questo vedo opportuno e possibile mettere in piedi un direttorio con Italia e Francia, poi Spagna e poi, forse, Benelux. Ma sapendo che la Germania sta lì, salda, per economia, per istituzioni, per partiti, nel cuore dell'Europa. È terra, è il solido. La Gran Bretagna è il mare, è il liquido; non a caso, l'isola se ne va per conto suo. Badate: terra e mare sono grandi categorie geopolitiche che dobbiamo imparare ad usare. Un'ultima, brevissima considerazione: Presidente, *historia magistra* ci insegna una cosa: non si unifica aspettando che le parti si mettano insieme. A parte l'eccezionalismo americano, un Paese senza storia statuale che confedera parti diverse (ma anche lì alla fine ci è voluto, a mezzo di guerra civile, un Nord che piega un Sud), l'Europa ci racconta altre vicende: in Italia c'è voluta la guida del Piemonte, in Germania la guida della Prussia. Senza i Cavour e i Bismarck non si fanno queste grandi cose. Il Presidente del Consiglio evoca spesso un'Italia alla guida dell'Europa. Realisticamente, non credo che possiamo pretenderlo. Se lanciamo l'idea della rimessa in marcia dell'Europa politica, possiamo ambire ad essere il primo vagone dopo la locomotiva. L'Italia è in posizione geopolitica quasi simile a quella della Germania: come la Germania sta strategicamente tra Est e Ovest, noi strategicamente stiamo tra Nord e Sud. Questa è la nostra specifica vocazione politica europea, che dobbiamo farci riconoscere, ma dobbiamo saperla praticare con abile intelligenza.

La mia generazione è cresciuta con il sogno di un'Europa finalmente unita, che metteva da parte i nazionalismi e abbatteva frontiere e permetteva così anche a quei popoli che erano stati divisi dalle guerre, come quello del Tirolo storico, di potersi ritrovare, in quella casa comune di valori a cui accennava anche il presidente Renzi. L'Europa o saprà mettere da parte gli egoismi nazionali o non ci sarà più. Il cambiamento che chiedono i cittadini europei vuol dire solo una cosa: mettere in campo politiche che aggrediscano la crisi economica. Occorre pertanto: riaprire una prospettiva di futuro, rimettendo in moto l'ascensore sociale; combattere le diseguaglianze e le ingiustizie sociali che in questi anni sono aumentate, ad iniziare dalla forbice nella distribuzione delle risorse e delle ricchezze e dare più fiducia ai territori e alle loro potenzialità. È questo il punto sul quale collassa tutto l'Occidente ed è qui che si afferma la spericolata idea del passato come di un tempo felice verso il quale è possibile ritornare. L'Europa, in questi anni, ha reso agli occhi dei cittadini una crisi di carattere finanziario, che andava perciò contrastata con politiche per la ripresa economica e non con le ricette dell'austerità, in una crisi della democrazia, della sua incapacità nel prendere le decisioni giuste rispetto alle paure, alle ansie, alle difficoltà delle persone. Guai a giudicare i cittadini che hanno votato per la Brexit, così come quelli che scelgono le forze antisistema. Il voto va accettato e rispettato, l'ha detto prima anche il Presidente, perché nell'antipolitica si nasconde la domanda di una politica migliore, più efficace nella sua azione, davvero in grado di migliorare la vita di tutti i giorni delle persone. Anche a Bruxelles, dove sono stato di recente per un incontro con i massimi vertici politici europei, ho capito che la più grande preoccupazione è l'affermazione del populismo e delle forze centripete, che in queste ore emergono anche in Francia e in Olanda. Bene. Cosa si aspetta ancora? Se si pensa di proteggere l'Europa sventolando i risultati delle borse o facendo parlare gli uomini della *City* si fa un errore clamoroso. La tecnocrazia e l'alta finanza sono il peggiore *spot* possibile per chi crede nel nostro Continente. Come autonomisti, abbiamo sempre sostenuto l'iniziativa del nostro Governo nei confronti dell'Europa. Governo italiano, lo ha detto oggi anche il Presidente del Consiglio, è stato tra i primi a evidenziare le contraddizioni e i problemi che sarebbero sorti se non si fosse cambiata strada. il ministro Padoan quanto dice che bisogna potenziare il piano Juncker per avere più investimenti e che bisogna costruire un meccanismo per gestire le fasi difficili e per non scaricare tutti i costi sui lavoratori, a condizione che sia solo il primo passo, Il contesto internazionale ci dice che senza l'Europa il mondo sarebbe ancora meno stabile. Ho partecipato, la settimana scorsa, al vertice NATO di Kiev dedicato alla questione ucraina. Ebbene, le tensioni di quell'area rischiano di divenire esplosive, l'assenza di dialogo tra le parti in gioco, la tentazione e la richiesta di una prova di forza, creano, giorno dopo giorno, i presupposti per rendere duratura l'instabilità dell'intera regione. Non oso immaginare cosa succederebbe se non ci fossero altre forze, come l'Europa o la NATO che, seppur con grande fatica e - fino adesso - scarsi risultati, non tenessero viva la fiammella di un possibile accordo per ristabilire la tregua in quell'area. Certamente l'accordo raggiunto tra Israele e Turchia è un segnale significativo in questa direzione ma quello ucraino, purtroppo, è solo uno dei tanti fronti d'instabilità e d'insicurezza del mondo. L'Europa, per essere autorevole, deve godere del sostegno dei suoi cittadini che si riconquista solo se riesce a trasmettere l'idea di un'istituzione vicina alle sofferenze, alle ansie e alle difficoltà di chi guarda il futuro come il tempo dell'incertezza. Credo che la sfida sia questa e vale a Roma, come a Londra, come a Madrid, come a Bruxelles, come a Washington. Siamo davanti a un passaggio epocale. Mai come ora dobbiamo esserne tutti all'altezza. Tutti noi dobbiamo avere consapevolezza di quanto è grande la posta in palio. L'Italia continui a fare la sua parte. Facciamo capire che non c'è più un solo minuto da perdere. *(Misto-Ipl)*. Signor Presidente, colleghi, non esagero nel dire che forse è uno dei momenti più difficili dal dopoguerra. Abbiamo legittimamente e responsabilmente paura perché sappiamo che il voto del Regno Unito potrebbe essere solo l'annuncio di ciò che può avvenire in ogni Paese Ci domandiamo: «Com'è possibile che il popolo britannico, conosciuto per la sua razionalità, abbia deciso di uscire?». Perché esiste una frattura; una frattura fra le *élite* e il popolo, fra le istituzioni e i cittadini e dunque anche fra l'Europa e le opinioni pubbliche nazionali. In più, l'effetto congiunto di crisi economica, migrazioni di massa e terrorismo ha creato nuove povertà, insicurezze, paure e dunque un sentimento diffuso di malessere. Oggi la vera sfida nel mondo è la capacità di far diventare la globalizzazione un fattore positivo di crescita per tutti e non, al contrario, un fattore negativo di squilibrio e di aumento della povertà. E solo con un'Europa unita si è in grado di affrontare una sfida del genere e di restare competitivi nel mercato internazionale a guida, ormai, di Cina e Stati Uniti. Da soli verremmo tagliati fuori da tutto. Cosa fare dunque adesso?

Il voto britannico è l'ultimo avviso per l'Europa e dunque è necessario rivedere subito la politica sociale ed economica dell'Europa; ma, allo stesso tempo, io dico, probabilmente in controtendenza al pensiero di molti, che il cambiamento deve partire da noi, dalla nostra mentalità che punta sempre il dito sempre verso gli altri e che alimenta le forze estremiste e illiberali che rischiano di portarci nel baratro. Il cambiamento deve partire dai singoli Stati membri, tutti, che devono mettere da parte gli egoismi. E, poi, diciamoci la verità: abbiamo sempre desiderato l'Europa, ma poi ne abbiamo sempre un po' diffidato. Infatti, finché non cederemo almeno parte delle sovranità nazionali, l'Europa esisterà solo nei nostri sogni. Finché non abbatteremo i muri nazionali, non ci sarà un'Europa più vicina ai suoi cittadini. La percepiremo come un'istituzione che si sovrappone a quelle nazionali, dunque raddoppiando le burocrazie In sostanza, occorre un'accelerazione dell'Unione politica, economica e bancaria. E io credo che se ciò non avverrà - e mi rendo conto che non sarà facile trovare il coraggio per fare questo salto - l'Europa sarà destinata a disintegrarsi, perché all'Europa o ci si crede o non ci si crede. Io ci credo. Il presidente Renzi ha detto che l'Europa è la nostra casa ed è vero: è la casa che ci ha permesso di migliorare la nostra vita e ci ha garantito la pace. Ma una casa va ristrutturata. Dunque il Presidente, domani, vada già con gli attrezzi per ristrutturarla, per ricostruirla. La situazione, lo sappiamo tutti, gli permette di imporre dei cambiamenti; lo deve fare con determinazione, con la sua determinazione, con la sua forza, per salvare questa Europa e la nostra casa.

Non penso che il Regolamento del Senato sia un bastione inespugnabile, Presidente. Potevamo tranquillamente decidere diversamente. Il Presidente del Consiglio avrebbe ascoltato quanto hanno da dire le opposizioni. Immagino che lo stesso arrivi in quest'Assemblea preparato, avendo condiviso con la propria maggioranza l'intervento di questa mattina. Abbiamo perso un'occasione; mi auguro che la prossima volta non accada. Mi posso anche permettere di dirle che l'avevo sentita in questi giorni: mi sembrava che fosse una mediazione ragionevole, nel momento in cui le forze di opposizione avevano anche ceduto al fatto di autoregolamentare il tempo. È quindi non senza difficoltà che in quest'Assemblea possiamo dedicare alcune brevi considerazioni al voto che ha destabilizzato l'Unione europea. Potrei indugiare nell'analisi del voto, delle sue cause, della sua matrice generazionale e declinazione territoriale, dei timori o, all'inverso, delle speranze di allargamento di un fronte antieuropeista; ma parlo in rappresentanza di una forza politica fortemente convita della necessità di salvare l'Unione europea, ma che, da tempi non sospetti, anche quando questo creava risolini Oltralpe e in Italia, è sempre stata molto critica nei confronti dell'austera euroburocrazia. Quindi ritengo che quest'ora che abbiamo a disposizione - devo dire, mal impiegata - debba essere finalizzata a sollecitare l'impegno del Presidente del Consiglio per i vertici che l'attendono questo pomeriggio e nei prossimi giorni; chiediamo fin d'ora

o l'Europa di Bruxelles è destinata ad avvitarsi su se stessa; vicina all'eurocrazia filotedesca, ma lontana, lontanissima, dai popoli europei. Non abbiamo più tempo: il Regno Unito, invece, non senza qualche pentimento, sembra voler prendere tempo: un tempo che i mercati non attendono per reagire. L'Italia paga più di altri, certamente più della Germania; le banche italiane sono le più danneggiate: si vendono BTP e si comprano *bond*. Il vertice a tre - non dimentichiamo che i *Premier* di Germania, Francia e Italia, più quello spagnolo, hanno la legittimazione politica di rappresentare il 70 per cento del prodotto interno lordo dell'Eurozona deve prendere misure e decisioni straordinarie, altrimenti si assumerà responsabilità straordinarie. oggi intende incalzare la cancelliera Merkel, da sempre restia a completare l'unione bancaria con la garanzia unica sui depositi? A rendere la BCE sempre più simile alla FED americana? A prevedere un vero piano di investimenti dopo il sostanziale fallimento del piano Juncker, che avrebbe dovuto rimettere in moto l'economia reale in molti Paesi europei e che invece ha prodotto soltanto effetti marginali, impercettibili?

L'Italia, ad esempio, ha tutti i requisiti per ospitare l'Autorità bancaria europea (EBA), come dice anche Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, e deve anche sforzarsi di attrarre i capitali, finora a Londra, che vorranno rimanere nell'Unione europea. Presidente del Consiglio, intende mantenere questo impegno? C'è, però, una domanda centrale alla quale vorremmo una risposta: essere l'Europa che vogliamo? Sarà forse quella in cui il forte *surplus* commerciale di Germania e Olanda sta creando danni immensi a tutto il resto d'Europa? A tal proposito voglio citare l'intervento dell'ex governatore di Bankitalia Fazio di qualche giorno fa. Diceva Fazio che se all'interno di uno stesso sistema c'è una parte dei partecipanti costretta a rimanere in equilibrio con i conti e a ridurre la spesa pubblica, e una parte invece sta in forte *surplus*, questa assorbe il risparmio del resto, creando deflazione. Il *surplus* della bilancia dei pagamenti di Germania e Olanda, con la Commissione che obbliga gli altri Paesi a stare in equilibrio, crea deflazione. l'Europa è quella in cui l'Italia si accontenta di trattare qualche zero, qualcosa di sforamento del rapporto tra *deficit* e PIL, mentre la Francia al G5 (che è un organismo nuovo, inedito, ma dove si discutono questioni vere e forse si prendono anche decisioni vere)

La Germania stessa è un problema per gli altri *partner* europei. Cito solo due esempi: i derivati ad orologeria che gravano sulle banche tedesche e il *surplus* delle partite correnti della bilancia dei pagamenti tedesca, che ha un effetto *killer*, ben maggiore dell'eccesso di *deficit* di altre economie del Continente.

La verità amara è che questa Europa fallimentare non ci prende sul serio. Non lo fa quando chiediamo l'abolizione delle sanzioni alla Russia, una delle scelte più miopi della politica internazionale dal dopoguerra. L'emergenza migranti nel Mediterraneo sembra sempre essere un problema nazionale e non comunitario: non può più essere quella di utilizzare la Marina italiana per soccorrere, molte volte a poche miglia dalle coste libiche, barconi in difficoltà e per raccogliere in mare uomini donne e bambini, a volte purtroppo già cadaveri. L'Europa avrà altro a cui pensare nei prossimi mesi. Ce la dovremo cavare da soli. Non dico di arrivare alla soluzione australiana, che con empirismo tipicamente anglosassone prende a traino con una fune i barconi e li riporta da dove sono partiti, spesso non importa nemmeno a quale costo di vite umane. Oggi più che mai occorre intervenire là dove si pone il problema con misure precise, radicali e chirurgiche. Abbiamo le professionalità per poterlo fare ed è solo un problema di volontà politica. Italia svegliati, l'Europa è distratta! Mi rivolgo al presidente Renzi, che in è in grado di ottenere un piano di investimenti europeo, anche attraverso eurobond, finalizzato al finanziamento degli strumenti necessari ad affrontare alla radice la catastrofe umanitaria nel Mediterraneo? passare finalmente alla fase tre di EUNAVFOR MED, come abbiamo accennato in precedenza? Di realizzare campi di accoglienza sulle coste nordafricane? Di concretizzare un piano Marshall per il Centro Africa, di cui abbiamo visto qualche timido accenno nel vertice de La Valletta del 2015, rimasto, come sempre in Europa, all'auspicio iniziale? Di ridare finalmente dignità e sicurezza al nostro Paese che, in piena allerta terrorismo internazionale, dimostra di avere delle frontiere colabrodo? Il *referendum* britannico è il principio della fine dell'Europa? È possibile. Di certo è la fine dell'Europa come l'abbiamo intesa fino ad oggi. Segna la fine dell'illusione che aggiustare l'edificio comunitario fosse questione di dettagli, di tecnicismi, di virgole da sistemare nelle infinite discussioni ai tavoli di Bruxelles.

Ma la preparazione e la traduzione di queste decisioni politiche nei *paper*, nei protocolli, nelle direttive e nei regolamenti è fatta dalla burocrazia europea: il livello politico deve dunque recuperare la responsabilità di ogni atto e di ogni decisione. Presidente Renzi, le chiediamo poche parole: oggi sono necessari fatti. Le chiediamo di non indugiare in *slogan* e frasi ad effetto. Le chiediamo di mettere da parte le sue ambizioni di *leader* politico e, anzi, di dimenticare anche il suo partito (cosa che, forse, fa anche volentieri). Lei oggi rappresenterà il Paese tutto, che ci piaccia o no, nel vertice più importante per il futuro dell'Europa. È tenuto dunque a prendere, davanti a questa Assemblea, il solenne impegno di far recuperare all'Italia il ruolo di motore di una nuova Unione, non più a trazione tedesca. Le democrazie europee alla fine degli anni Trenta non avevano voglia di morire per Danzica. Sicuro che la Germania della cancelliera Merkel non possa essere finalmente ricondotta a ragione, prima che qualcuno parli, con qualche ragione, di quarto Reich? un'Unione che si occupi più dei popoli che delle regole, più di educazione, ricerca e investimenti, più della disoccupazione e della povertà e meno dei pochi decimali nel rapporto tra *deficit* e PIL. È necessaria un'Europa della pace, anche economica. La aspettiamo al suo rientro, signor Presidente del Consiglio. Questa Assemblea non le farà sconti: non può farlo, per i cittadini che rappresenta, per il Paese tutto, per l'Europa in cui abbiamo creduto e in cui vogliamo ancora credere per i nostri figli.

i Gruppi di maggioranza hanno ceduto i loro tempi all'opposizione. Questo è potuto avvenire perché si era già a conoscenza del fatto che i tempi dell'intervento del Presidente del Consiglio sarebbero stati ristretti, presupposto che noi non potevamo conoscere se non dopo che si è verificato; in ogni caso, inoltre, c'è stato un accordo tra i Gruppi e non un intervento del Presidente. Questo per la precisione.

riflessioni proposte dal senatore Tronti, abbiamo ascoltato solo contributi critici alla proposta e all'iniziativa del Governo, quindi credo che il Presidente del Consiglio abbia sin dall'inizio potuto raccogliere elementi e certamente altri ne avrebbe potuti raccogliere. *(Commenti).* È stato amaro, molto amaro, signor Presidente, il risveglio di venerdì scorso dopo che eravamo andati tutti a letto tirando un sospiro di sollievo alle prime notizie sull'esito del *referendum*, notizie poi totalmente smentite dal risultato finale. Vorrei subito dire, perché non è stato sottolineato fino ad ora, che sono comunque importanti le rassicurazioni ascoltate in queste ore circa il fatto che il nostro Paese corre rischi molto contenuti e che comunque sono già predisposte eventuali iniziative per fronteggiare le conseguenze finanziarie. Tuttavia, comunque la si pensi, credo non sia esagerato definire Brexit un punto di svolta di portata storica per tutti i Paesi europei e non soltanto per l'Europa. Vorrei dire al senatore Lucidi che il problema non è il non voler prendere atto della volontà popolare, tutt'altro. Noi abbiamo preso atto - eccome - di quella volontà; semmai il problema è che oggi dobbiamo essere tutti consapevoli di essere di fronte a un bivio sarà decisivo quale delle due strade di questo bivio noi sceglieremo per incamminarci nei prossimi mesi. Sarà una scelta decisiva per il futuro delle nostre società non credo sia esagerato dire che sarà decisivo per i futuri equilibri mondiali. Non è un caso che, subito dopo quel risultato,

non è un caso che il tema Brexit sia entrato a tutto tondo e prepotentemente nella campagna elettorale che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Si è ampiamente detto e scritto sulle ragioni di quel risultato; anche oggi abbiamo sentito parlare della parte incompiuta del lavoro di costruzione dell'Unione, di tutti i rischi che sono di fronte a noi. Non voglio ripetere cose note e in gran parte condivisibili e devo confessare un certo fastidio anche nel riascoltare il solito *refrain*, sentito ogni qual volta si è registrato un passaggio difficile nella storia europea. Penso da ultimo a quello che accompagnò la discussione dopo il rischio Grexit, anche se mai prima d'ora l'Europa si era trovata di fronte a una crisi di questa portata. Già da qualche anno, nonostante le sempre più significative avvisaglie circa la seria difficoltà del rapporto tra le istituzioni europee e le opinioni pubbliche nazionali, nazionali, ascoltiamo solenni proclami a cui, puntualmente, non sono mai seguiti i concreti cambiamenti necessari.

poi durante il semestre europeo a guida italiana e, infine, nei tanti, forse troppi vertici europei in cui si è cercato di convincere con insistenza gli altri Paesi a cambiare rotta, ad agire più che a dichiarare a condividere la gestione dei *dossier* più significativi su cui misurare la capacità e - vorrei dire - l'utilità dell'Europa. Vorrei anche aggiungere

Caro senatore Centinaio, altro che traghetti per clandestini: le nostre missioni internazionali in mare hanno saputo coniugare un'opera di polizia con un'azione umanitaria che fa onore al nostro Paese. Anche grazie a tutto questo, oggi il nostro Paese è chiamato oggettivamente a svolgere un ruolo di *leadership* per superare questa crisi, a iniziare dall'incontro in programma questa sera a Berlino. Nei tanti commenti al voto è stato molto frequente il richiamo all'immigrazione come fattore che, più di ogni altro, avrebbe determinato quel comportamento elettorale. In realtà, da troppo tempo gli immigrati si sono di fatto trasformati nel capro espiatorio perfetto in cui il rancore di segmenti di opinione pubblica si è progressivamente canalizzato.

avranno sempre più mano libera quegli imprenditori del malessere, così solerti e in azione nelle ultime ore nell'alimentare quell'utopia stregata contro l'Europa. La stessa domanda di sicurezza, che è forse una delle più forti nelle nostre società, oggi può essere seriamente soddisfatta soltanto in una dimensione europea. modo, l'Europa deve mettere i Governi in condizione di sviluppare quelle politiche di investimento che aiutano a creare lavoro e a ridurre diseguaglianze sociali non più sopportabili. se non si agisce subito in questa direzione, la breccia aperta dalla Brexit diventerà una grande falla e sempre più rischia di concretizzarsi quel terribile presagio che un uomo attento come Soros ha segnalato avantieri in un suo editoriale parlando di una possibile disintegrazione europea.

e l'instabilità, profondamente legati tra loro perché, in un circolo vizioso, l'uno alimenta l'altro. Il populismo, che ormai si è accampato in quell'incrocio dove si incontrano la solitudine e la ribellione, ha bisogno si nutre di sistemi politici e istituzionali instabili e, per questo, fragili e incapaci di decidere. Dopo la Brexit è preoccupante che in un grande Paese come la Spagna si siano svolte due elezioni in sei mesi

perché è la stabilità la condizione per agire e battere il populismo; e anche di qui passa la tenuta e lo sviluppo di una prospettiva europea. è il momento della verità per il progetto europeo. Si è detto che l'Europa resta la nostra casa, che bisogna ristrutturarla, ma soprattutto che bisogna agire concretamente e subito. Su questo crediamo valga la pena insistere nel vertice di questa sera e nel successivo Consiglio europeo. In momenti come questi, il Capo di un Governo dovrebbe poter contare sulla solidarietà di tutto il Parlamento di tutte le forze politiche, perché è in gioco molto di più di qualche voto. Certamente questa sera e domani il Governo potrà contare sul convinto consenso del nostro Gruppo.

Capisco le sue preoccupazioni, senatore Paolo Romani, ma è prematuro stabilire già oggi che mancano questi fondi, anche se lei sa benissimo che l'Italia ne è il principale utilizzatore. Noi siamo d'accordo a rafforzare il piano Juncker, ma dare queste cifre come

No a qualsiasi rinnovamento automatico delle sanzioni, ma necessità di portare ogni volta la discussione a livello politico. Se il senatore Paolo Romani e gli altri firmatari sono d'accordo con queste riformulazioni, il parere del Governo diventa favorevole. PRESIDENTE.

Presidente, le riformulazioni del Governo non sono per noi accettabili, perché essenzialmente viene esclusa in maniera a questo punto evidente il CETA come atto atto di competenza del Parlamento italiano. Il CETA, per chi non lo sapesse, è un accordo simile al TTIP, ma che in questo caso riguarda

dall'avere voce in capitolo sui trattati che riguardano la vita, il futuro e il destino non solo dell'economia, ma del modo di vivere delle persone. Ricordo infine al Ricordo infine al sottosegretario Gozi che nella Conferenza tenutasi tra i Presidenti dei Parlamenti nazionali dello scorso anno, proprio qui a Roma, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera si espressero nella stessa identica maniera, insieme ai loro omologhi degli altri Paesi, chiedendo l'impegno dei Governi affinché tutti i trattati, compreso il CETA, fossero sottoposti comunque al vaglio dei Parlamenti nazionali. Questo significa inevitabilmente una discordanza, ma la cosa che ci preoccupa molto più è che ci sia una volontà esplicita di sottrarre ai cittadini la scelta finale sul proprio destino.

accettabili e accessibili da parte nostra, non c'è chiarezza invece sulla questione inerente a EUNAVFOR MED. Noi riteniamo che la fase 2 debba assolutamente concludersi: non possiamo più consentire che la Marina italiana vada a prendersi migliaia di persone direttamente quasi sulle coste libiche. Pertanto, è necessario dare un segnale forte di sospensione di tale attività, non volendo determinare nel Mediterraneo un cimitero

Presidente, se le altre riformulazioni sono accettate dal senatore Paolo Romani, se questo è l'unico punto

Governo, onorevoli colleghi, da troppo tempo nella politica europea sono venuti meno quella visione utopica e quello slancio ideale dei padri fondatori. Il vuoto emotivo lasciato dal venir meno del coraggio e dell'utopia europeista europeista è stato progressivamente riempito dalla paura e dalla diffidenza nei confronti di istituzioni ritenute troppo distanti e straniere. Sull'Europa, come fosse un untore manzoniano, si è riversata la frustrazione degli emarginati della globalizzazione, si è scatenata la paura dell'immigrazione incontrollata, si è concentrato il rancore dei disillusi, la rabbia della periferia contro il centro. Tutto questo è stato reso possibile anche dalla codardia di una classe politica europea che ha trovato comodo scaricare sull'Europa le responsabilità di scelte, tanto necessarie quanto impopolari. *Leader* piccoli piccoli hanno lasciato che l'Europa fosse il capro espiatorio di ciò che andava male. Sarebbe assurdo, quindi, oggi pensare che si possa salvare l'Europa trovando un nuovo capro espiatorio, magari proprio lo strumento referendario o rallegrarsi perché in Italia non è possibile indire un *referendum* come quello britannico. Questo modo di pensare non salverà l'Europa, perché l'Europa si salva e progredisce se un'ampia maggioranza di cittadini europei condivide e legittima il processo d'integrazione europeo. Esiste un problema democratico in Europa ma non è rappresentato dal rischio di nuovi *referendum*. È la mancanza di legittimazione democratica delle scelte nevralgiche che l'Europa ha preso e che la crisi economica ha messo in luce in maniera drammatica. Agli occhi di tutti noi europei, oggi, oggi, chi decide le sorti della Grecia? Il Parlamento europeo o la cancelliera tedesca? Con quale diritto, e con quale legittimazione? Quale dibattito pubblico ha accompagnato il *fiscal compact*? Quale dibattito pubblico è previsto per il TTIP? Che ruolo hanno avuto i cittadini europei nel trattare le condizioni alla Grecia o all'Italia? Con quali strumenti è sanzionabile democraticamente il responsabile di questo disastro? La crisi politica dell'Europa non è causata dal *referendum* britannico. La crisi politica dell'Europa è causata dai suoi *leader* che continuano ad ignorare la gravità di queste semplici domande. E alla crisi democratica si è accompagnata in questi ultimi anni una crisi culturale e sociale. sociale. Come pretendere che le classi medie impoverite dei Paesi ricchi d'Europa siano ben disposte ad essere solidali nei confronti dei popoli degli altri Stati dell'Unione più in difficoltà, dopo decenni di politiche neoliberiste che hanno abituato a considerare la solidarietà e la giustizia sociale come concetti antiquati e pericolosi, ostacoli allo sviluppo economico? Mai come oggi è evidente come per salvare l'Europa sia necessario un processo di integrazione meno timido e più profondo, che consenta all'Unione di dotarsi degli strumenti di cui ha bisogno per dare le risposte che i cittadini si aspettano. I problemi della democrazia si risolvono con più democrazia. I problemi di integrazione con più integrazione. L'Italia, come Paese fondatore dell'Unione, deve portare avanti e proporre con coraggio un percorso costituente per un'Unione europea diversa e compiutamente politica. Si colga da questo momento di crisi l'occasione per il necessario passo in avanti verso gli Stati Uniti d'Europa, per cambiare rotta alle politiche economiche dell'Unione e correggere quelle regole stupide che hanno senso solo laddove si voglia continuare a privilegiare alcuni Stati a spese di altri. L'Italia abbia il coraggio e la lungimiranza dei padri fondatori e riassuma quel ruolo politico centrale che ha sempre avuto nella storia del nostro Continente. Le risoluzioni presentate sono molte e varie. Il Governo ha dato l'assenso solamente ad alcune, e la contrarietà a quella presentata dal Gruppo SEL e Sinistra Italiana, che io ho sottoscritto

Signor Presidente, abbiamo ascoltato come sempre le belle parole del Presidente del Consiglio. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni che ho annotato: dopo la Brexit non possiamo far finta di niente; il voto democratico non va ignorato; abbiamo portato il nostro contributo perché qualcosa cambiasse; l'Europa deve combattere una battaglia di giustizia sociale; manca consapevolezza della gravità della situazione. Infine, l'ultima dichiarazione del Presidente del Consiglio è stata: l'Europa deve smuoversi.

non possiamo che prendere atto che alle parole non segue una presa di coscienza rispetto alle vere necessità che devono essere portate avanti da parte del nostro Governo. Nel recente *forum* economico di San Pietroburgo il presidente Renzi a parole, a favore della revisione delle decisioni assunte in materia di sanzioni contro la Russia. Fin dal primo momento la Lega Nord ha affermato con forza che le sanzioni sono una vera e propria follia, hanno provocato danni incalcolabili alla nostra economia e nessun risultato diplomatico positivo. Le sanzioni non vanno prorogate, ma annullate. C'è un'unica verità, purtroppo: l'Europa non ha a cuore il benessere dei propri popoli, delle proprie comunità e dei propri cittadini. Abbiamo chiesto al Governo di assumere una posizione ferma e chiara, non ambigua. Le belle parole e le buone intenzioni non bastano più. I segnali di sfiducia e l'insofferenza dei popoli europei sono sempre più evidenti. La Brexit insegna: il rischio che la dissoluzione europea diventi una valanga inarrestabile è un rischio reale. Il Governo, esprimendo contrarietà alle nostre risoluzioni, non evidenzia una presa di coscienza responsabile di ciò che sta accadendo, non mostra la volontà di cambiare, ma di perseverare nelle attuali politiche europee dettate da un *establishment* lontano anni luce dalle necessità dei cittadini europei. Questa è l'Europa di chi porta avanti gli interessi di pochi contro gli interessi dei molti, è una follia che voi appoggiate e sostenete servilmente e che ci porterà a un futuro fatto di disoccupazione di massa, di di sempre maggior diseguaglianza sociale, di povertà e di miseria. Questa, signor Presidente, non è la nostra Europa. Non è l'Europa che vogliamo,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i risultati del *referendum* britannico hanno determinato una svolta profonda negli assetti complessivi della politica, in Gran Bretagna innanzitutto, dove si è aperta una crisi i cui sbocchi sono, al momento indefinibili. Sullo sfondo è infatti il problema della stessa unità politica del Regno Unito. Cosa farà la Scozia? E che processi scatteranno in Irlanda, i cui passati conflitti sanguinosi avevano conosciuto una loro ricomposizione solo in nome dell'Europa? Questo per non parlare della prospettiva economica di quel Paese, la cui potenza, soprattutto finanziaria, era garantita dalla relativa solidità della sterlina e dalla capacità del suo doppio ancoraggio all'euro e al dollaro. La City rimarrà la grande piazza finanziaria che conosciamo o sarà insidiata da Milano, come ha proposto il sindaco Sala? E come si comporteranno Parigi e Francoforte, le grandi multinazionali, il domicilio fiscale di FCA? Rimarrà ancora la terra d'Inghilterra? Ma se Atene piange, Sparta non ride. Sarà pur vero che il colpo nei confronti dell'Europa avrà un impatto minore, ma sarà pur sempre un colpo, non tanto sul piano economico e finanziario - ci sarà anche quello - ma dal punto di vista politico, soprattutto geopolitico. Non dimentichiamo, infatti, che a seguito di Brexit le distanze tra Parigi e Mosca sono diminuite e non a vantaggio dell'Unione. è poi il rischio di un effetto domino che può portare da un lato all'uscita di altri Paesi, dall'altro ad accentuare quella frattura che all'interno degli stessi Paesi fondatori divide le forze riformiste da quelle populiste. Comunque la si metta, quindi, il 23 giugno non sarà ricordato come una giornata da festeggiare. E per favore risparmiateci la retorica del trionfo della democrazia. Una decisione di tale portata è stata avallata da un voto minoritario che ha riguardato più o meno un terzo degli aventi diritto. Episodio analogo a quanto è avvenuto in molti Comuni italiani, con Sindaci eletti da una minoranza, meno del 25 per cento del corpo elettorale. Ed allora consentitemi di richiamare l'antica lezione di Rousseau e lanciare un grido d'allarme sul pericolo delle manipolazioni dei sistemi elettorali rispetto al necessario manifestarsi di quella volontà generale che è, questa sì, il fondamento vero di ogni democrazia. Ma noi siamo italiani, portatori di una cultura che ci consente di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, e quindi di scorgere anche nei momenti più difficili un sottile filo di speranza a cui appellarci nell'idea che non tutto il male viene sempre per nuocere. Ed allora, ecco che a guardare oltre la brutta congiuntura di questi giorni, Brexit non ha fatto altro che confermare che eravamo nel giusto quando indicavamo i pericoli e le miopie di *élite* dirigenti troppo chiuse in una prospettiva nazionale di breve periodo. Oggi far finta che nulla sia avvenuto sarebbe solo un suicidio annunciato. Dobbiamo, invece, cambiare e cambiare in fretta per recuperare il tempo perduto. Nella nostra risoluzione abbiamo accennato ai principali *dossier*: migrazione, sviluppo, investimenti. La declinazione tecnica di una svolta che presuppone la progressiva costruzione di una volontà comune. Non abbiamo bisogno di muri per frenare la libera circolazione degli uomini, ma questi stessi muri non questi stessi muri non possono esistere per le politiche di bilancio, per gli assetti finanziari o per le regole bancarie. Pur con la necessaria gradualità, da una dimensione puramente nazionale, occorre inseguire un respiro sempre più comunitario. Questo è l'invito che rivolgiamo al presidente Renzi, nel momento in cui si appresta a manifestare la posizione dell'Italia, nei prossimi vertici. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che dietro Brexit c'è anche il fallimento dì un asse politico - quello franco-tedesco che aveva l'ambizione di guidare l'Europa verso un radioso avvenire ed invece si è risolto in una grave sconfitta, alla quale si deve rimediare. Ma per ottenere un risultato credibile è necessario che gli stessi protagonisti del passato abbiano la forza di rigenerarsi aprendosi agli apporti che possono venire da uomini di buona volontà che hanno solo a cuore una storia, quella europea, che non consideriamo assolutamente finita.

del Regno Unito dall'Unione europea. E purtroppo ciò condizionerà i lavori di domani e dopodomani. Purtroppo l'eventualità oggi è divenuta certezza: il Regno Unito ha democraticamente scelto di uscire. Stiamo assistendo, all'indomani del responso della consultazione, a cosa sta accadendo nei mercati, anche oggi, ed alle conseguenze negative e pesanti per l'Unione europea e per lo stesso Regno Unito, che rischia di implodere (basta vedere cosa sta accadendo in Scozia e in Irlanda), che non sono oggi totalmente calcolabili ma solo ipotizzabili. È certo però che il filo comune che lega tutti i commenti sul tema è l'affermazione che l'Unione europea è stata percepita, in particolare dai britannici, in particolare dai britannici, come un'organizzazione vincolante per certi aspetti e incapace di risolvere tempestivamente le questioni emergenti di rilevanza sociale come un presunto afflusso di immigrati alle sue frontiere (faccio presente che quando si parla di immigrati nel Regno Unito si considerano immigrati anche gli stessi italiani e tutti coloro che arrivano dal Continente) e soprattutto la crisi economica e finanziaria che ha investito in questi anni l'intero mondo e rispetto alla quale, anche grazie agli interventi della BCE, siamo riusciti a contenerne i danni. Non si può negare che questa sia la vera difficoltà e non è tanto l'Europa, in quanto progetto costitutivo, ma piuttosto gli Stati nazionali, che non sono in grado, da un lato, di far fronte da soli ai processi di globalizzazione, di condividere la loro sovranità su tematiche fondamentali, come l'emigrazione, la lotta al terrorismo o la gestione delle crisi finanziarie, per riuscire a far svolgere all'Europa il ruolo che le spetta nel sistema mondiale. Ciò è tanto più vero nel caso del Regno Unito che, geloso della propria assoluta sovranità decisionale, si è sempre mantenuto ai margini dell'Unione europea, opponendosi a ogni ulteriore integrazione, di fatto limitando la possibilità per l'Unione europea di rafforzare il suo quadro istituzionale ed offrendo linfa alla crescita nel proprio Paese di posizioni euroscettiche e perfino anti-europee. anche le recenti concessioni strappate da Cameron non hanno fatto altro che alimentare e accentuare l'estraneità del Regno Unito (non a caso lo stesso Cameron si è giocato il suo stesso futuro politico). Del resto nel Regno Unito il dibattito sulla convenienza di partecipare o no alla Unione europea ha radici lontane: era già vivo ai tempi dei Trattati di Roma. Ci troviamo quindi ad affrontare un periodo molto complesso, un periodo nel quale è necessario assumere decisioni rapide e immediatamente praticabili sui grandi temi che da tempo sono sul tavolo: il tema della migrazione, il tema dell'occupazione, della crescita, degli investimenti per cercare di ridurre al massimo i disagi derivanti dall'abbandono dell'Unione europea da parte del Regno Unito, ma soprattutto per dare risposte ai bisogni dei cittadini del resto dell'Unione. A nostro parere, quindi, è essenziale che, fin da oggi, nell'incontro cui il presidente Renzi parteciperà, si diano dei segnali significativi, che possano proseguire nei due giorni successivi. A nostro parere, ad esempio, sarebbe importante rivedere e dare maggiori poteri al Parlamento europeo. Può essere questa l'occasione propizia per rivedere anche i vincoli e le regole del Patto di stabilità e del *fiscal compact*. Una riflessione che deve fare necessariamente tesoro di quanto successo il 23 giugno. In tema di investimenti pubblici e privati sarà bene immaginare un meccanismo che consenta di non considerare ai fini dei bilanci nazionali gli investimenti destinati ad infrastrutture, che sono quelli maggiormente destinati a produrre occupazione. Può essere l'occasione per definire uno schema di assicurazione europea contro la disoccupazione, proposto dal ministro Padoan. Insomma, la risoluzione sottoposta al nostro esame cerca di affrontare tutti questi problemi,

cercando di superare le secche che molto spesso hanno frenato il compimento di politiche efficaci e danno un'immagine di un'Europa spesso lenta e inconcludente, lontana dalla vita dei cittadini. Particolare attenzione deve essere posta alla capacità dell'Europa di dare risposte pronte ai problemi emergenti, come le crisi migratorie ed economiche, rispetto ai quali le soluzioni danno l'idea di essere lontane o, addirittura, producono effetti deleteri, come si è visto nelle nelle reazioni elettorali nei vari Paesi. Basti vedere la Spagna, che alla fine rimane in una situazione di grande precarietà. A questo proposito ci auguriamo, quindi, che la proposta italiana sul *migration compact,* che ridisegna le politiche europee per quanto riguarda i rapporti con i Paesi terzi e, in particolare, con i Paesi africani, sia finalmente approvata. Essa rappresenta un contributo decisivo alla strategia dell'Unione europea per il contenimento dei flussi migratori. L'azione che sta portando avanti il Governo è assolutamente coerente con lo spirito e la lettera dei Trattati fondativi; uno spirito che, però, deve essere ritrovato e rinnovato e che, a nostro avviso, deve avviarsi ad un parziale superamento dei temi riguardanti l'unione economica economica e commerciale dovendo guardare di più alla solidarietà e sussidiarietà, che sono la linfa della coesione e alimentano la partecipazione reale degli Stati a questa istituzione.

Noi dobbiamo riprendere il concetto di Europa, quell'Europa in cui crediamo, quell'Europa che desideriamo: «Perché alla fine dei conti svegliarsi per l'Europa significa semplicemente tornare se stessa: una terra che ha scelto la pace perché i suoi padri avevano conosciuto la guerra. Che ha investito sulla crescita perché i suoi padri avevano conosciuto la fame. Che costruisce i ponti perché sa quanto male hanno fatto i muri. E che deve riprendersi gli ideali, non solo i parametri e i vincoli». del Consiglio, che queste parole la guidino nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, perché in questo momento ha una responsabilità grande, non solo per il nostro Paese, ma per l'intero Continente.

avanzato un invito ad andare oltre una discussione e delle proposte puramente retoriche e a entrare nel merito di alcune proposte secche, che avanziamo nella proposta di risoluzione

un sussidio europeo di disoccupazione e, soprattutto, il finanziamento di un piano serio - e non quello di Juncker - di investimenti pubblici, anche con la possibilità di emettere eurobond. La citata risoluzione

Le cause che hanno portato al risultato del *referendum* sono molteplici e tutt'altro che scontate. L'onda lunga della crisi globale, il persistere di situazioni di crisi, con la conseguente constatazione che il livello di benessere diminuisce e che le disparità tra le classi sociali crescono, è alla base dei fenomeni di scetticismo nei confronti dell'Europa e, più in generale, nei confronti della politica tradizionale, che imperversano nel nostro Continente. C'è poi la scarsa consapevolezza dei veri rischi che vengono da Sud, da Est e, nel prossimo futuro, da Nord, accerchiando letteralmente il vecchio Continente, sotto la pressione di terrorismi e migrazioni epocali. La paura dell'immigrazione è una questione che, fino a questo momento, non è stata ben gestita dalla Unione europea. Il cittadino britannico ha probabilmente pensato che, chiudendosi a riccio, avrebbe evitato questi rischi, dimenticando che le leggi britanniche sono le più sciaguratamente permissive e hanno consentito lo stabilirsi di *enclave* dove il radicalismo islamico ha prosperato e prospera. la superficialità del dibattito nel corso della campagna referendaria, basato quasi interamente sull'istintività e sullo scontro e pochissimo sulla razionalità: si tratta di una responsabilità grave, che va attribuita anzitutto alla *leadership* politica dei conservatori, che non ha saputo spiegare le vere ragioni del *remain*. Quali sono le strade da seguire per permettere al progetto europeo di continuare? Non tentare di tornare indietro. Ciascun popolo si assume le proprie responsabilità e ne deve pagare le conseguenze. ripartire da tre. Serve una Europa a tre: la prima fu quella dei Padri fondatori, la seconda quella dell'attuale allargamento e il processo deve essere condotto dai tre attori che, attraverso i loro grandi uomini, furono protagonisti dell'idea fondativa: Germania, Italia e Francia, che però devono rifarsi ai valori di Adenauer, De Gasperi e Schuman. Occorre riscrivere la Costituzione europea, a partire da una chiara affermazione delle radici storiche, culturali e religiose del Vecchio continente, dando spazio, anche linguistico, alle diverse tradizioni e dando, ad esempio, un ruolo di primo piano anche all'italiano e allo spagnolo a fianco del francese, dell'inglese e del tedesco, e avere come obiettivo la crescita del benessere di tutti, non di alcuni a spese di altri. Bisogna superare gli egoismi nazionali o particolari, che ci farebbero ridurre l'Europa a un'articolazione di piccole Province, consegnandoci nelle mani del potente di turno: Russia, Cina, Islam, ma anche gli stessi Stati Uniti. Prevedere flessibilità e non rigidità burocratiche. Qui la responsabilità è fortemente nelle mani della Germania, ma gli altri - noi compresi - non possono scaricare le colpe sui tedeschi, ma devono pretendere rispetto a tutti i livelli: politico, economico, sociale, culturale. Attuare con coraggio politiche di sviluppo, per aumentare il benessere individuale e collettivo. Finora - diciamolo pure - il solo Mario Draghi è parso avere una lucida strategia in questa direzione, ma da solo non può pensare di reggere, anche perché le misure economico-finanziarie, se non hanno alle spalle una solida comune visione politica, rischiano di fallire miseramente. Ricomporre le divisioni, muovendosi in una logica di inclusione: popolari, socialisti e liberali devono convincersi a governare insieme ovunque, almeno per i prossimi dieci anni, per portare il Continente fuori dalla crisi e per riguadagnare il consenso dei cittadini verso la politica, battendo demagogie e qualunquismi. Siamo di fronte a processi lunghi, difficili, ma la via è una sola e senza ritorno. Auguriamo a noi stessi di saper rispondere a queste sfide per non consegnare alle future generazioni un Continente peggiore. Valutiamo l'ipotesi di introdurre l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea per colmare il distacco tra i cittadini e l'Unione europea. Variamo un grande piano di investimenti (con o senza eurobond), ben oltre quello finora adottato da Juncker, per favorire l'occupazione, la crescita, il benessere, l'eguaglianza. Completiamo l'unione bancaria con la garanzia unica sui depositi: un progetto concreto per fronteggiare la disoccupazione giovanile. Mettiamo in atto il *migration compact* e la strategia globale di politica estera, già proposti dall'Italia. Quali sono stati, signor Presidente, i limiti di fondo della costruzione europea? L'euro è una moneta senza Stato. È stato scisso, cioè, il legame storicamente sempre esistente fra moneta e autorità statale, che esercita la propria sovranità tramite il fisco e la moneta. Occorre rapidamente superare questa contraddizione di fondo; il paradosso di una politica di forte austerità realizzata proprio durante la più lunga e grave recessione del dopoguerra. Si è così calpestato, e letteralmente rovesciato, ogni insegnamento di Keynes, che assegnava al saldo di bilancio una funzione anti-ciclica e non pro-ciclica. Certamente, occorre impedire i disavanzi di bilancio negli anni di espansione dell'economia, ma imporre vigorose politiche di riduzione del disavanzo, in una fase economica fortemente recessiva, ha solo prodotto milioni di disoccupati. Occorre adesso riflettere su un'Europa diversa, ma sarebbe un errore desistere dal progetto di integrazione comunitaria. Al contrario, è necessario porsi in sintonia con un orizzonte strategico che preveda un incremento delle politiche comuni, una politica della difesa, una politica estera, una politica delle sicurezza e, in prospettiva, anche una politica economica comune. L'Europa deve darsi un volto nuovo, che stimoli e dia rilancio all'economia e che ci faccia sentire meno soli e più forti. Che il futuro debba seguire questa direzione emerge anche dalla constatazione che il 75 per cento dei giovani britannici ha votato per il *remain*: chi ha sperimentato direttamente le opportunità che l'Europa offre, da queste opportunità non vuole recedere. Il progetto degli Stati Uniti d'Europa, il progetto dei Padri fondatori, che lo concepirono in un momento di maggiori difficoltà rispetto a quelle odierne, va ripreso e attualizzato. Per rilanciare il processo di integrazione comunitaria, allora, occorrerà riflettere sugli errori commessi. Ogni ragionamento su un nuovo inizio assumerebbe in effetti i contorni del vano esercizio accademico, se non partissimo dal dato di fatto che l'Unione europea a guida tedesca ha adottato in questi anni, nel contesto di una recessione più grave di quella del '29, politiche economiche orientate all'assoluta austerità, le quali, sommate a emergenze senza precedenti come quelle rappresentate dalla decomposizione geopolitica e dai flussi migratori che ne sono derivati, hanno finito per dare fiato al populismo e al razzismo. È nostro compito impegnarci attivamente nel cambiare l'Europa contribuendo a renderla più umana, più giusta, più vicina ai cittadini, più coesa e fortemente radicata nei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Dobbiamo contribuire attivamente al rafforzamento della solidarietà e della coesione all'interno dell'Unione, in un momento - diciamolo pure - molto difficile dove siamo chiamati ad affrontare sfide enormi che toccano da vicino la vita dei cittadini. Queste sfide richiedono una vera politica economica comune basata su crescita e occupazione, e una politica migratoria comune che sia efficace e di lungo termine. L'Europa è la nostra casa - condivido il pensiero del Presidente del Consiglio - la casa di tutti noi. Impegniamoci a migliorarla e a renderla garanzia per le nuove generazioni.

quindi suppongo che non sia neanche stata letta ed è stata rifiutata semplicemente perché è del Movimento 5 Stelle, che in questo momento non è troppo popolare.

alla permanenza forzata dell'Italia nell'euro, abbiamo proposto un *referendum* consultivo per chiedere agli italiani cosa pensano dell'eurozona e non abbiamo mai messo in discussione l'importanza della costruzione di un'Unione europea basata sul sogno dei Padri fondatori; pensiamo quindi ad un'Unione europea dell'accoglienza, ad un'Unione europea della democrazia, dove il Parlamento

grazie a tutto

è quella che vuole il Movimento 5 Stelle. Su questo non desidero dilungarmi, perché tanto anche questo viaggio del presidente Renzi è quasi privo di senso nel momento in cui l'Europa sta crollando. Il senatore Monti a suo tempo disse che quello che stavano costruendo i Paesi era una polvere d'Europa, un'Europa che non aveva più ragion di essere così come era e questo è diventato una realtà.

non lottiamo affinché vadano in un Paese piuttosto che in un altro, ma affinché ci siano regole chiare, affinché chi ha diritto possa rimanere e chi non ha diritto venga rimandato nel proprio Paese; questa però deve essere una gestione europea e non dei singoli Paesi. Voteremo invece a favore della proposta di risoluzione n. 2, che parla delle sanzioni alla Russia. Anche questo è un argomento che abbiamo sollevato varie volte in numerose interrogazioni. Le sanzioni alla Russia sono ridicole, danneggiano l'Italia, servono solo a inginocchiarsi di fronte agli Stati Uniti d'America e a creare un polo che escluda la Russia.

in attesa di un *welfare* condiviso in Europa, siamo d'accordo che ognuno debba poter gestire il proprio Stato con le deroghe riconosciute alla Gran Bretagna.

siamo costretti ad andare a leggere le pagine del TTIP in camere segrete, privi di telefonino e con tempi contingentati, senza la possibilità di fare delle fotocopie. C'è il segreto di Stato sulla gestione delle regole fitosanitarie di un Paese.

a cominciare a confrontarvi anche con le opposizioni sui temi europei, perché l'Europa è di tutti.

agli interventi dei singoli, che possono avere un peso limitato. Ma così va. Del resto, Renzi non ascolta neanche Putin e nessun altro. Renzi può ascoltare chi vuole, tanto sbaglierebbe comunque.

I problemi sono già tanti e un'Europa spezzettata nei singoli Stati sarebbe ancora più facilmente fagocitata da capitali che non vengono più solo dai luoghi dove storicamente si formano, ma anche dall'Oriente o dal Sud del Pianeta. Quindi noi

grazie a tutto Quando nel 2011 cadde il Governo guidato da Berlusconi, denunciammo la miopia dell'Europa e il contrasto, non a caso, con Merkel e Sarkozy. Anche la nostra appartenenza al Partito popolare europeo non è un'appartenenza subalterna, ma siamo carichi di storia, di valori e di tradizioni

che il nostro documento pone, riguarda la politica internazionale. Il Governo Berlusconi apparteneva saldamente al PPE e all'Europa, ma con una presenza dialettica e non subordinata, soprattutto rispetto ai voleri e agli strapoteri della Germania, alle manovre speculative e a tutto quello che poi è successo e che non dimentichiamo, dalla vendita dei titoli italiani a tutto ciò che poi si è verificato. Ma ricordo anche che quel Governo fu capace di aprire ad un dialogo sempre migliore e più proficuo con la Russia. Noi prendiamo atto del fatto che le nostre valutazioni sono state in parte condivise dal Governo, ma riteniamo che l'Unione europea, che continua a sanzionare in maniera negativa la Russia, stia creando un danno alle nostre imprese. Vorrei anche dire a Renzi - glielo dico a futura memoria - che inutile che vada a San Pietroburgo a dire che si riaprono i canali di dialogo con la Russia di Putin, se poi, poche ore dopo, conferma il rinnovo delle sanzioni per altri mesi, con l'entusiastica adesione dell'Italia. Si vede che, giocando con il telefonino, non ascoltava quello che Putin gli diceva durante quel *summit*. Anche su questo rivendichiamo la strategia dei Governi del passato, come sul tema dell'immigrazione. Il Governo Berlusconi veniva preso in giro per il dialogo con Gheddafi. Ebbene, in quella fase però le partenze venivano bloccate dalla Libia. Abbiamo sopportato qualche bizzarria di Gheddafi. Poi, l'Occidente ha proclamato la guerra, per volontà - guarda un po' - di Cameron, che si deve dimettere, di Sarkozy, che fu sconfitto, di Obama e della Clinton, il primo che sta per lasciare la Presidenza e la seconda che speriamo non ci arrivi. Con quella guerra, vinta dall'Occidente, abbiamo causato quel disastro libico che non si sa dove andrà a parare. Noi facemmo una politica di realismo, che riuscì a contenere i flussi incontrastati di immigrazione. non è che siamo europeisti teorici, ma siamo europeisti con una posizione autonoma, da protagonisti, che ci ha portato spesso anche a scontri nell'ambito dell'Unione europea. Qualcuno fu contento di quelle difficoltà e di quelle manovre? Ebbene, avevamo ragione noi ed avevano torto quelli che spalleggiavano

in Spagna. Mi segnala una collega che nessuno del Governo ci ascolta; ma questo è normale. A forza di non ascoltare, lascerete i banchi del Governo; lo sappiamo, non c'è dubbio. Per quanto riguarda EUNAVFOR MED, il Governo ha accettato la nostra stesura. Lo dico al ministro Pinotti, visto che ha competenza operativa. Ricordatevi di quello che avete accolto. alla fase 3, quella con la collaborazione del Governo libico per combattere davvero gli scafisti, o si può attuare rapidamente in un tempo ragionevole, oppure va sospesa la missione. Un conto è il soccorso umanitario, un altro conto è mettere nel Mediterraneo decine di navi che sono un'istigazione agli scafisti ad attuare i loro traffici: questo sta accadendo. Tra venerdì e domenica, signori del Governo, sono stati portati in Italia 12.000 clandestini, e non erano tutti donne e bambini; il telegiornale inquadra giustamente la donna incinta che commuove tutti o il bambino, ma il 90 per cento era composto da giovani solidi e robusti, che poi in Italia si lamentano se non c'è il *wi-fi* in albergo,

*(PD)*. Signor Presidente, sono tra quanti ritengono che grandi questioni che mettono in gioco trattati internazionali molto complessi, che per decenni hanno dispiegato già i loro effetti, non dovrebbero poter essere sottoposte a *referendum*, e con lungimiranza la nostra Costituzione non consente che i trattati internazionali vengano sottoposti a *referendum*. la ragione si capisce: il *referendum*, per sua natura, semplifica i problemi sino a radicalizzarli e può produrre conseguenze anche non volute persino da chi lo ha promosso. Pensavo che nel Regno Unito avrebbe vinto il *remain* e che le immaginabili conseguenze disastrose del *leave* lo avrebbero fatto perdere. Viceversa, le cose sono andate come sappiamo. Chi crede e rispetta le regole della democrazia deve ora accettare senza indugi il risultato del voto, cercare di comprenderne le ragioni, lavorare per capire dove abbiamo sbagliato anche noi e cosa dobbiamo fare per affrontare una condizione europea che è diventata molto difficile. se l'Italia, come deve e può fare, vuole contribuire a far volgere in positivo questa nuova e grave crisi europea, deve chiedere che le procedure di uscita

dentro per i vantaggi che offre la grande economia dell'Unione e fuori perché non piace collaborare all'accoglienza dei migranti. L'Europa deve tanto al Regno per la forza con cui ha resistito al nazismo ed ha consentito a tutti noi un futuro democratico e libero. Il Regno Unito è e deve Non è certo l'amicizia tra l'Europa e il Regno Unito ad essere in gioco. Ma non è questo il tempo né dei temporeggiamenti né delle concessioni o degli statuti speciali di privilegio. La volontà che i cittadini britannici hanno manifestato è quella di uscire dall'Unione e l'Europa ha il dovere di rispettarla pienamente, senza compromessi e ancor meno senza pasticci. Anche noi vediamo i pericoli e i rischi di un'Europa burocratizzata e lontana dai bisogni umani e sociali dei suoi cittadini, lontana dalla cultura e dalle tradizioni dei popoli che la abitano. Ma noi crediamo che l'idea di Europa sia molto più forte dei suoi malanni e vogliamo aiutarla a correggersi. Noi sappiamo che nel tempo della globalizzazione, della più avanzata rivoluzione tecnologica della storia, delle migrazioni di interi popoli, il destino nostro e dei nostri figli è strettamente legato alla capacità di far crescere l'Europa, non alle manovre per farla crollare. Diverso è il giudizio politico nei confronti della *leadership* britannica che, senza considerarne appieno le conseguenze, questo *referendum* ha prima evocato e poi cercato, coltivato, sino a farlo celebrare e, infine, a perderlo. Nessuno dei grandi *leader* che in passato hanno governato il Regno Unito, da Churchill a Macmillan e alla Thatcher, avrebbe mai consentito che venisse messa a rischio la sopravvivenza dell'Unione europea con tanta leggerezza. In molti Paesi dell'Unione sono presenti forze politiche che pongono al primo posto del loro programma la morte dell'euro e la disgregazione dell'Unione, che vogliono far fare a tutti noi un passo indietro di 70 anni. È questa l'ideologia di fondo che ha prevalso nel *referendum* britannico, incurante non solo del futuro dell'Europa, ma anche della stessa integrità del Regno Unito dove, visto l'esito del *referendum*, è possibile si riaprano sia la questione irlandese, sia il delicatissimo nodo della indipendenza scozzese. Lo chiamano effetto domino. Le forze politiche democratiche europee debbono fare tutto il possibile per impedire che si allarghi una regressione di molte decine di anni e per fermare un processo fatto di spinte alla frammentazione, di eccesso di nazionalismi e localismi, di egoismi politici e, soprattutto, di vista corta, molto corta. Nessuna nazione europea, nemmeno la ricca Germania, è in grado, da sola, fuori dall'Unione, di fronteggiare le sfide del nostro tempo. A prescindere dalle conseguenze che avrà in termini economici, industriali, di integrazione e persino militari, l'uscita del Regno Unito pone i popoli e i Parlamenti europei di fronte alle loro responsabilità storiche, politiche e morali. Un grande quotidiano italiano nelle edizioni di sabato, ha riassunto le nostre responsabilità con un titolo a caratteri cubitali: «Europa, svegliati».

di rango europeo. Non possiamo più continuare a declamare con retorica che vogliamo più Europa, senza dire contemporaneamente cosa in concreto significhi più Europa, quali sono le strade che vogliamo percorrere per ottenerla e i tempi che ci servono per completare l'opera, quali sono i prezzi da pagare in termini di sovranità nazionale, quali i ritorni in termini di sicurezza economica e strategica del continente. Più Europa vuol dire principalmente più democrazia e più politica. Per avere più democrazia serve un Parlamento europeo più forte. Non è difficile, ma bisogna volerlo. Per avere più politica serve lavorare per un'Europa federale alla quale gli Stati, anche sacrificando parte consistenti della loro sovranità, affidino sicurezza, difesa e politica estera, bilancio e fisco. che si assuma la responsabilità della lotta al terrorismo internazionale, delle politiche delle migrazioni e delle politiche di sviluppo e di espansione. Non serve a nessuno un'Europa burocratica che pretenda di misurare i millimetri delle vongole, che contesti la produzione del formaggio di fossa, che disquisisca di agriturismi e persino di rosmarino, come ieri, ironicamente, ha detto in un'intervista Romano Prodi. Ai 500 milioni di cittadini europei serve un'Europa che si ispiri ai principi dei Padri fondatori e che si impegni a risolvere in primo luogo, prioritariamente, i grandi problemi geopolitici, economici e sociali del nostro continente e non dia, invece, prevalenza a una minuziosa ed eccessiva attività regolatoria in questioni che converrebbe lasciare alla disciplina degli Stati nazionali. Le senatrici e i senatori del Partito Democratico apprezzano e sostengono la linea politica che il nostro Governo e il Presidente del Consiglio stanno tenendo in Europa e considerano con favore il rispetto con cui le posizioni italiane vengono accolte. A cominciare dalla richiesta di maggiore attenzione alle politiche di sviluppo e alla sollecitazione per un drastico cambio di rotta, che sappia dare un respiro di lungo periodo alla politica europea dell'immigrazione. Oggi l'Italia è ascoltata in Europa non solo per la qualità delle misure che propone, ma anche per la stabilità politica che da qualche anno esprime. In un contesto internazionale dove si formano parti considerevoli dei destini delle nazioni, veniamo tutti pesati per la stabilità che riusciamo a esprimere e per la responsabilità delle nostre posizioni. Nel giorno in cui l'esito del voto spagnolo non risolve l'incertezza del quadro politico di quel Paese, guardiamo la carta dell'Europa e osserviamo la stabilità molto precaria di tante nazioni indebolite da difficili condizioni politiche, dalla crisi economica, dal ritardo delle riforme, grazie a tutto con un avanzato e significativo programma di riforme, rispettoso dei parametri di Maastricht. Da qui viene il credito internazionale di cui godiamo, che ci consente di portare con autorevolezza all'attenzione dei *partner* europei ed extraeuropei la nostra visione dell'Europa e i nostri interessi nazionali. Ad una crisi economica ormai decennale, con le sue drammatiche conseguenze sul piano sociale, alle migrazioni di massa, alle numerose e pericolose tensioni internazionali, si aggiungono ora gli effetti gravi della Brexit. Dico alle forze politiche di maggioranza e di opposizione: difendiamo la stabilità del nostro Paese, non sciupiamola per le nostre beghe interne. Ricordiamoci che la stabilità avvantaggia tutti, mentre l'instabilità danneggia fortemente anche chi la determina.*(Applausi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

Grazie.